Signor Presidente, Governo, colleghi, nel presente decreto-legge, recante un complesso di misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, si nota un apprezzabile cambio di paradigma rispetto al passato, sia per quanto concerne la tecnica di scrittura legislativa, caratterizzata da concretezza, sia per una più immediata comprensione delle nuove disposizioni. Il provvedimento riflette una chiara visione riformista, interessando quattro aree di intervento di assoluta profondità sociale, ed è per questo che è stato oggetto di una profonda analisi, con ampio spazio alle audizioni di tutte le parti sociali interessate e una completa e vivace discussione in Commissione. La prima area di intervento dà seguito alle previsioni della legge di bilancio per il 2023. Quest'ultima ha prospettato un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, stabilendo, nelle more della riforma ora definita dal presente decreto, sia l'abrogazione dell'istituto del reddito di cittadinanza, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sia una revisione della disciplina di tale istituto per il 2023. In primo luogo, con gli articoli da 1 a 11 del presente decreto si istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, spettante in favore dei nuclei familiari in cui vi sia almeno un soggetto minorenne o avente almeno sessanta anni di età o disabile - come aggiunto in sede referente, ampliando la platea - almeno un componente in condizione di svantaggio inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali. Riguardo ai disabili, si fa riferimento alle categorie di disabilità poste dalla disciplina regolamentata in materia di ISEE. In sede referente sono stati inoltre attenzionati i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alle violenze di genere, specificando che costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini ISEE. In merito agli ulteriori requisiti soggettivi o inerenti al nucleo familiare, di cui all'articolo 2, si rileva in primo luogo che quelli inerenti alla cittadinanza, alla residenza o al soggiorno del richiedente il beneficio in oggetto sono analoghi a quelli già previsti per il reddito di cittadinanza. Si segnala che viene operata una riduzione da dieci a cinque anni del requisito di durata minima della residenza in Italia nel periodo di vita precedente alla domanda del beneficio, ferma restando la condizione della residenza continuativa in Italia negli ultimi due anni precedenti alla domanda. A quest'ultimo riguardo, il comma 10 introduce una definizione specifica di continuità di residenza. I requisiti inerenti alle condizioni economiche del nucleo familiare, concernenti sia i valori massimi dell'ISEE, del reddito familiare, del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, sia l'assenza di godimento di alcuni beni durevoli particolari, sono analoghi a quelli previsti per il reddito di cittadinanza. Tra le differenze si segnala che il limite relativo al reddito familiare è parametrato in base a una scala di equivalenza. La misura del beneficio economico in oggetto è determinata nell'articolo 3, modificando quelli previsti per il reddito di cittadinanza. Una prima differenza consiste nell'applicazione di un nuovo parametro moltiplicativo in ragione della diversa scala di equivalenza summenzionata. Una sostanziale differenza deriva dal diverso regime di durata e di rinnovo, in quanto per l'assegno di inclusione, dopo i primi diciotto mesi, il rinnovo è ammesso il rinnovo è ammesso per dodici mesi (anziché diciotto), ferma restando la sospensione di un mese dell'erogazione del beneficio prima di ogni rinnovo. L'articolo 4 del decreto concerne in primo luogo la procedura per la domanda e per il riconoscimento del beneficio economico in oggetto. La domanda è presentata all'INPS, anche tramite gli istituti di patronato e di assistenza sociale e - come aggiunto in 10a Commissione - tramite i centri di assistenza fiscale conosciuti come CAF. Il riconoscimento della misura presuppone la sottoscrizione da parte del richiedente di un patto di attivazione digitale. Quest'ultimo deve essere sottoscritto in una piattaforma digitale del sistema informativo per l'inclusione sociale lavorativa (SIISL). Alla sottoscrizione del suddetto patto conseguono, da un lato, il riconoscimento dell'assegno di inclusione nel mese successivo, dall'altro lato, l'applicazione di ulteriori procedure e obblighi. L'inadempimento di tali obblighi determina la decadenza del beneficio ai sensi dell'articolo 8. In particolare si prevede che i servizi sociali effettuino una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare intesa alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Nell'ambito di tale valutazione i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni, attivabili al lavoro, vengono avviati ai centri per l'impiego

da parte dei componenti del nucleo familiare maggiorenni o di età inferiore ai sessanta anni, che esercitino la responsabilità genitoriale, non occupati, non frequentanti un regolare corso di studi, né titolari di una pensione diretta e che non abbiano determinate cariche di cura relative a figli o familiari disabili. Sono esclusi da tali obblighi le persone affette da patologia oncologica, i soggetti con disabilità rientranti nell'ambito di applicazione del cosiddetto collocamento obbligatorio nonché, come aggiunto in sede referente, i soggetti inseriti nei percorsi di protezione e di fuoriuscita dalle violenze di genere. In ogni caso i soggetti esclusi dai suddetti obblighi possono richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento al servizio personalizzato. Riguardo il sopramenzionato patto di servizio personalizzato le Regioni possono prevedere che la sottoscrizione e la relativa presa in carico siano effettuate anche presso i soggetti accreditati per i servizi per il lavoro. Seguirà un decreto ministeriale proprio per individuare le misure per il coinvolgimento dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e la formazione. I commi dal 9 all'11 dell'articolo 6, parzialmente riformulati in sede referente, disciplinano l'utilizzo per il potenziamento degli interventi dei servizi sociali di risorse finanziarie già stanziate. Riguardo alla modalità di erogazione l'articolo 4, al comma 8, prevede che l'assegno di inclusione sia corrisposto mediante uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato carta di inclusione, utilizzabile per acquisto o, entro i limiti previsti dal medesimo comma, per prelievi di contante. Si esclude che la carta possa essere utilizzata per giochi che prevedono vincite di denaro o altre utilità. Inoltre, come definito in 10a Commissione, la carta non può essere utilizzata per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici o di prodotti alcolici. L'articolo 7, nel quale in sede referente sono state inserite alcune modifiche tecniche, individua le amministrazioni e le autorità competenti per i controlli dell'assegno di inclusione. Ad esso occorre aggiungere i Comuni che sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici. L'articolo 7 interessa anche i criteri e le modalità di acquisizione dei dati

nonché per alcune fattispecie di falso o di omissione nelle comunicazioni o dichiarazioni e per il rifiuto di un'offerta di lavoro subordinato rientrante nell'ambito della fattispecie di cui al successivo articolo 9. Quest'ultimo, nel testo parzialmente riformulato in sede referente, distingue a seconda che l'offerta di lavoro sia a tempo indeterminato o a termine e, nell'ambito della prima tipologia contrattuale, disciplina distintamente l'ipotesi in cui nel nucleo familiare vi siano figli di età inferiore a In 10a Commissione si è inserita al lato degli 80 km la percorrenza in massimo centoventi minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 9 prevede che l'assegno sia sospeso in caso di rapporto di lavoro a termine di durata compresa tra uno e sei mesi. L'erogazione del beneficio riprende al termine del rapporto. Il periodo di durata di quest'ultimo e il reddito da esso derivante non rilevano ai fini dell'applicazione dell'assegno. L'articolo 10 prevede una serie di incentivi per l'assunzione di soggetti beneficiari dell'assegno per l'inclusione nonché una prestazione aggiuntiva per i beneficiari

con riferimento alle assunzioni in oggetto effettuate a seguito di loro specifica attività di mediazione; un incentivo per alcuni enti e imprese, con riferimento alle assunzioni in oggetto relative a persone con disabilità ed effettuate a seguito di attività di mediazione da parte dei medesimi enti o imprese. La summenzionata prestazione aggiuntiva per i beneficiari dell'Assegno di inclusione è riconosciuta in un'unica soluzione ed è pari a sei mensilità dell'Assegno di inclusione (calcolate nel rispetto di un limite pari a 500 euro mensili). L'articolo 11 prevede un'attività di monitoraggio e di valutazione relativi all'attuazione dell'Assegno di inclusione nonché l'istituzione di un Osservatorio sulle

inserito in sede referente in 10a Commissione - reca, con riferimento all'intero decreto-legge, una clausola di salvaguardia relativa alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano; lo stesso articolo reca, con riferimento alle suddette Province autonome, clausole specifiche, relative all'Assegno di inclusione o a misure analoghe. L'articolo 13 reca disposizioni transitorie, di coordinamento e finanziarie. Si rileva, in primo luogo, che il comma 3 reca un intervento di coordinamento al fine di assicurare l'inclusione nel regime sanzionatorio previsto per il Reddito di cittadinanza anche degli illeciti in materia commessi nella fase finale di applicazione dell'istituto. La novella di cui al successivo comma 6 conferma che alle categorie di soggetti rientranti, dal 1° gennaio 2024, nell'ambito dell'Assegno di inclusione continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2023 il Reddito di cittadinanza senza l'applicazione del limite di sette mensilità introdotto dalla legge di bilancio per il 2023. Il comma 5 inserisce un'ulteriore fattispecie per la quale si esclude tale limite; nuova norma, come parzialmente riformulata in sede referente, fa riferimento ai soggetti che, entro il 31 ottobre 2023, siano stati presi in carico - in quanto non attivabili al lavoro - dai servizi sociali. Passando al secondo Capo del provvedimento, l'articolo 14 - il cui testo è stato integrato in sede referente - reca un complesso di modifiche alla disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le modifiche concernono, tra gli altri, profili attinenti al medico competente, alle attrezzature di lavoro, agli edifici scolastici. L'articolo 15 prevede che, per le finalità ivi indicate, gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongano con l'Ispettorato nazionale del lavoro, con conseguente messa a disposizione delle stesse anche in favore del Corpo della Guardia di finanza, così come riformulato in Commissione. L'articolo 16 prevede che

dal presente articolo un'omologa previsione, relativa alle Province autonome di Trento e di Bolzano. I commi 1 e 2 dell'articolo 17 istituiscono un Fondo per il riconoscimento di una misura di sostegno economico in favore dei familiari degli studenti, ivi compresi quelli universitari o dei percorsi di istruzione e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative. La definizione dei requisiti e dei criteri di determinazione della misura di sostegno, nonché delle modalità di accesso al Fondo, è demandata a un decreto ministeriale. I successivi commi 4 e 5 - parzialmente modificati in sede referente - recano alcune integrazioni alla disciplina sui percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Le novelle riguardano, tra l'altro, il principio della coerenza dei suddetti percorsi con il piano triennale dell'offerta formativa

della formazione aziendale. In base a tale estensione, le categorie di soggetti analiticamente individuati dal comma 2 - operanti nei suddetti settori come docenti o con altre funzioni o ivi attivi come studenti o allievi - sono comprese nel regime assicurativo. L'articolo 19 prevede un incremento della dotazione del Fondo nuove competenze, mediante l'impiego di risorse relative al periodo 2021-2027. Con le risorse del fondo sono finanziati parte della retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate ai percorsi formativi. L'articolo 20 prevede la possibilità di accoglimento di alcune domande relative alla misura di sostegno economico in favore degli utenti dei servizi di trasporto cosiddetto *bonus* trasporti). L'articolo 21 consente che alcune risorse previste per la formazione professionale ed eventualmente non utilizzate siano destinate a progetti rientranti in programmi gestiti dall'ANPAL. L'articolo 22 modifica la disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico. La novella concerne la maggiorazione specifica dell'assegno attribuita per i casi in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro e il valore dell'ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari ad un determinato limite. Al riguardo giova evidenziare che la finalità della misura è incentivare l'occupazione dei genitori che fanno parte del medesimo nucleo famigliare. L'articolo 23 modifica la disciplina delle sanzioni penali o amministrative pecuniarie per l'omissione del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale da parte dei datori di lavoro, nonché da parte dei committenti dei contratti di co.co.co. rientranti nella cosiddetta gestione separata dell'INPS. L'articolo 23-*bis* - inserito in sede referente - introduce la possibilità di versamento della contribuzione pensionistica in relazione ad alcune fattispecie di avvenuto annullamento automatico - in seguito a norme speciali - dei debiti contributivi. L'articolo 24 - ampiamente riformulato e integrato in sede referente - modifica, in primo luogo, la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato. Vengono ridefiniti i presupposti di ammissibilità (cosiddette causali) di una durata dei contratti superiore a dodici mesi e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi. La nuova disciplina, oltre a confermare che la causale può consistere in esigenze di sostituzione di altri lavoratori, reinserisce la causale costituita da fattispecie previste dai contratti collettivi, riproponendo a regime una norma transitoria, operante fino al 30 settembre 2022; sopprime sia la causale di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, sia la causale di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria; introduce la causale - applicabile solo con atti stipulati entro il 30 aprile 2024 e solo in assenza delle suddette previsioni da parte dei contratti collettivi applicati in azienda. Viene inoltre modificata la disciplina dell'applicazione delle causali - come ora ridefinite - relativamente alle proroghe e ai rinnovi dei contratti di lavoro a termine.

lavoro a tempo indeterminato. L'articolo 25 modifica la disciplina dell'istituto transitorio dei contratti di espansione, la cui finalità è di consentire un ricambio generazionale nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese. L'articolo 26 reca semplificazioni in merito agli obblighi di informazione e di pubblicazione, relativi al rapporto di lavoro, che devono essere adempiuti dal datore di lavoro o dal committente in favore dei lavoratori. L'articolo 27 riconosce un incentivo ai datori di lavoro privati per le nuove assunzioni, effettuate nel periodo 1° giugno 2023-31 dicembre 2023, a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, di giovani al di sotto dei trenta Tale incentivo è concesso per un periodo di dodici mesi e nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. L'articolo 28 prevede un incentivo all'assunzione, da parte di enti del terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni. L'articolo 29 modifica la disciplina del trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti dagli enti del terzo settore. In sede referente l'articolo è stato riformulato e si sono altresì introdotte novelle corrispondenti nella disciplina specifica relativa alla impresa sociale. L'articolo 30 prevede una possibile fattispecie di prolungamento - non oltre il 31 dicembre 2023 - del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga esplicita ai limiti di durata stabiliti dalla disciplina relativa al suddetto trattamento. L'articolo 31 reca alcune disposizioni per il completamento dell'attività di liquidazione della compagnia aerea Alitalia. L'articolo 32 prevede, per il 2023, un incremento delle risorse per il finanziamento statale delle convenzioni tra l'INPS e i CAF. L'articolo 33 dispone un finanziamento straordinario in favore dell'Agenzia industrie difesa.

per il periodo 1° luglio 2023-31 dicembre 2023, incrementa di quattro punti percentuali la misura della riduzione temporanea, già prevista per il 2023, dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate fasce di L'articolo 39-*bis,* inserito in 10a Commissione, riconosce, al fine di garantire a stabilità occupazionale e di sopperire alla eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale in via transitoria, ovvero dal 1° giugno al 30 settembre, un trattamento integrativo riconosciuto dal sostituto d'imposta.

(*fringe benefit*). Tale regime transitorio più favorevole è riconosciuto ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. In sede referente, è stato approvato un elevamento della stima del relativo onere finanziario, al fine di tener conto degli effetti dell'esenzione anche sulla base imponibile della contribuzione previdenziale. L'articolo 41 incrementa il Fondo per la riduzione della pressione fiscale nella misura di 4.064 milioni di euro per il 2024. L'articolo 42 istituisce un fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro per il 2023, per le attività socio-educative in favore dei minori; il fondo è destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, intese al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri svolgenti attività educative e ricreative. In sede referente, è stata poi inserita una proroga fino al 31 dicembre 2023 di alcune disposizioni in materia di lavoro agile (*smart working*), per il settore del lavoro privato, relative in particolare a genitori

dell'apposito elenco ISTAT, siano considerati nel calcolo del reddito assoggettato al limite massimo retributivo per i lavoratori pubblici. Introduce alcuni obiettivi da perseguire in materia di politica di remunerazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei suoi diritti di azionista di società. L'articolo 44 concerne la quantificazione e la copertura degli oneri di cui al presente decreto-legge e reca alcune clausole contabili, rimodula la misura dell'aliquota dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio delle imprese assicurative, ed infine, incrementa il Fondo rotativo del Mediocredito centrale per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese nella misura di 545 milioni di euro per il 2023.

anche a una parte politica del nostro Paese, che invece ha suscitato numerose polemiche che in questa sede non voglio assolutamente ricalcare. Desidero invece

Si tratta quindi di un provvedimento che vede il Governo confrontarsi con queste sfide economiche che sono ardue per il Paese, perché parlare di politiche del lavoro non è mai semplice, non lo è mai

produttivi del nostro Paese e di offrire sostegno alle imprese e ai consumi, a chi realmente oggi è impedito a svolgere anche un'attività lavorativa. È evidente quindi che in questa congiuntura molto delicata

evitando sprechi, soprattutto in misure che sono puramente assistenziali; alleggerire gli oneri delle imprese, in modo da liberare risorse che servono per gli investimenti; favorire così a livello individuale un reddito aggregato, quel sostegno ai consumi che oggi è la base dell'economia. Quindi, in un momento anche economicamente particolare e difficile a causa dell'inflazione, abbiamo la necessità di dare più soldi, più ricchezza alle nostre famiglie e sostenere i consumi. Il decreto lavoro ha puntato su questi due aspetti fondamentali. Abbiamo introdotto l'assegno di inclusione, che va a sostituire il famigerato reddito di cittadinanza, e abbiamo continuato a

dell'esame che c'è stato in Commissione, sono stati numerosi i provvedimenti e soprattutto gli emendamenti accolti che sono stati proposti dal Gruppo parlamentare di Forza Italia. Cito, a titolo di esempio, l'ampliamento della platea dei destinatari degli interventi di inclusione sociale, finanziati attraverso il fondo povertà, includendo anche quelle persone e famiglie che, pur in condizioni di estrema povertà, certificata dai competenti servizi sociali dei Comuni, mancano dei requisiti per beneficiare di tali misure e degli interventi ad esse connessi. È prevista una maggiore rappresentanza dell'Arma dei carabinieri nell'Ispettorato nazionale del lavoro, proprio in tema di controlli nel settore del lavoro. Sono stati poi accolti anche alcuni nostri ordini del giorno, importanti e vincolanti, anche per programmare altri interventi legislativi interventi legislativi da parte del Governo, per estendere l'applicazione dei *fringe benefit* aziendali ai lavoratori, per rimodulare l'importo delle pensioni minime e soprattutto l'importo delle pensioni di invalidità, che vanno aumentate. Questo è un aspetto politico importante.

delle persone tra i diciotto e i cinquantanove anni; l'assegno viene erogato dal 2024 a coloro che hanno un reddito inferiore a 9.360 euro, limite che scende per quelle famiglie che sono composte da *over* 67 o disabili. Al limite, si sommano ulteriori 3.360 euro per l'affitto. Fino a dicembre 2023 si prosegue quindi con il reddito di cittadinanza. Il meccanismo di assegnazione del nuovo assegno passa anche attraverso l'INPS. L'assegno vale 500 euro ed è erogato per diciotto mesi per i nuclei familiari con disabili e *over* sessantenni. Come noto, noi abbiamo sempre avuto una posizione a favore

il sostegno alle fasce più deboli con reddito più basso delle famiglie andasse sempre sostenuto. Quindi, il Governo oggi va in quella direzione. Solo negli anni 2020 e 2021 i dati che sono stati raccolti, anche in tema di reddito di cittadinanza usato male, quindi rispetto alle cosiddette truffe che sono state certificate, le prestazioni erogate non dovute sono state pari a circa 200 milioni di euro, cioè il triplo di quanto riscontrato nel 2020. Sono continuate anche in questi anni le truffe sul reddito di cittadinanza: una situazione inaccettabile che andava necessariamente arginata. Pertanto, i requisiti sono stati oggi modificati per accedere all'assegno, ma ipotizzando che ci sarà ancora chi proverà ad accedere al nuovo beneficio pur non avendone le caratteristiche. Sono state quindi previste, nel decreto lavoro, delle sanzioni più pesanti, che prevedono la reclusione fino a sei anni per chi rilascia dichiarazioni false. Sono previsti quindi filtri ulteriori, non solo al momento della richiesta dell'assegno, ma anche per il mantenimento dello stesso, prevedendo la verifica sulle banche dati dei requisiti per poterne godere. È previsto uno sgravio contributivo fino a 8.000 euro per i datori di lavoro che assumono il

oggi un ulteriore taglio di 4 miliardi di euro a favore dei redditi bassi, quindi fino a 35.000 euro. Per la copertura si utilizza tutto l'indebitamento che abbiamo approvato, pari a 3,5 miliardi di euro nell'ultimo DEF 2023, ai quali poi si aggiungono anche altre variazioni di bilancio. Il taglio è complessivamente, in questo questo anno, tra la manovra finanziaria di dicembre e l'ulteriore taglio con il DEF, di 7 punti percentuali sui redditi fino a 25.000 euro, il che significa che si può arrivare fino a 100 euro in più in busta paga. Fino a 35.000 euro il vantaggio fiscale è complessivamente pari a 6 punti percentuali. Anche questa battaglia sul cuneo fiscale ci appartiene da sempre e ora più che mai, per incrementare il reddito reale delle famiglie e limitare soprattutto la rincorsa tra salari e prezzi. La scommessa, da qui alla prossima legge di bilancio di dicembre, è quella di trovare le coperture adatte a rendere strutturale la misura del cuneo

a restituire anche un valore al reddito delle nostre famiglie, che dobbiamo impegnarci tutti, con questo Governo e in questa legislatura, a rendere strutturali.

Governo, cittadini in ascolto, devo dire che sono veramente colpita dall'indifferenza di questa maggioranza per le vere istanze del Paese. Indifferenza e non solo, perché in questi otto mesi di governo avete più volte dimostrato, a noi nelle Aule e agli italiani che tutti i giorni vivono i problemi reali, che siete totalmente sordi alle difficoltà delle persone, manifestando addirittura arroganza e totale mancanza di rispetto per chi ha bisogno di uno Stato veramente solidale e vicino ai più deboli. Questo decreto-legge che dovremmo chiamare "precariato", che il Governo ha beffardamente chiamato decreto lavoro, è forse l'emblema più alto dell'irriverenza mista ad arroganza con cui state continuando a tutelare i forti, facendo cassa su chi è in ginocchio e non ce la fa più. Il nostro non è un Paese per giovani e non lo è sempre più per colpa di questo Governo. Dopo aver detto ai nostri ragazzi di essere degli scansafatiche, dei "divanisti", dei fannulloni, dei parassiti, dopo aver detto loro che devono smettere di sognare il lavoro e la professione per cui hanno studiato tanto, con grandi sacrifici delle famiglie che li sostengono, magari mandandoli a studiare fuori sede nelle università più accreditate, per dar loro un'opportunità in più di trovare il lavoro, dopo aver fatto credere loro che il Governo avrebbe contrastato la denatalità, con interventi a sostegno delle famiglie e dei giovani, che la loro famiglia sognano di metterla su, avete sfoderato un decreto che spegne con ferocia le speranze di un futuro dignitoso per intere generazioni, condannandole al precariato selvaggio. precariato selvaggio, fatto di contratti a tempo determinato e *voucher* come regola e non come eccezione, contratti che ai nostri giovani non permettono nemmeno di comprare un frullatore a rate, figurarsi di ottenere un mutuo e di poter mettere su famiglia. Contratti che agevolano solo chi mette il profitto davanti a tutto, davanti alla dignità delle persone, alle loro storie, quelle che sabato scorso abbiamo portato in strada a Roma, in piazza, ma che volutamente fate finta di non ascoltare. Accanto a questi giovani che il lavoro lo cercano, nel giorno della festa del lavoro avete conciato per le feste anche chi già lavora e che, nonostante abbia un impiego, non arriva a fine mese.

Non arrivano a fine mese quei 5 milioni di lavoratori e lavoratrici che, pur spaccandosi la schiena quaranta ore a settimana, hanno una paga da 4-5 euro lordi l'ora da contratto collettivo nazionale, avete capito bene. Sto parlando di persone in carne e ossa, che devono scegliere, se fare la spesa e far mangiare i loro figli o curarsi e comprare le medicine. In tema di lavoro sottopagato devo purtroppo ritornare ai nostri giovani, perché questo riguarda anche i più brillanti, che sono costretti a lasciare l'Italia, la famiglia, le persone care perché, facendo lo stesso lavoro all'estero, guadagnano in media il 40 per cento in più. Come ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, andare all'estero deve essere una scelta, ma non obbligata. A ciò avete associato lo smantellamento dell'unica vera misura di protezione sociale esistente in Italia, percepita - pensate un po' - anche da 200.000 lavoratori poveri. Sto parlando ovviamente del reddito di cittadinanza, che con questo provvedimento avete provato maldestramente a copiare, il tutto solo per far cassa. Secondo uno studio di Etica ed Economia, con il passaggio dal reddito all'assegno di inclusione, la spesa annua si ridurrà di circa 3,5 miliardi e il risparmio più consistente riguarderà i nuclei con un unico componente. Ma un significativo risparmio di spesa peserà su tutte le dimensioni familiari, mentre si continuano a stanziare risorse per l'industria delle armi - complimenti - come avete fatto anche con questo decreto. *(Applausi)*. Si tagliano fondi per il contrasto alla povertà in un momento in cui l'inflazione resta al 7 Per quanto riguarda invece i cosiddetti occupabili, nel testo del provvedimento in esame il Governo è riuscito addirittura a scrivere che il percettore del supporto per la formazione e il lavoro - ricordo, sono appena 350 euro al mese può autonomamente individuare progetti di formazione. Ciò significa che, ancora una volta, tradite una promessa elettorale, quella mai mantenuta di far partire da gennaio 2023 i famosi corsi di formazione e ciò perché in questi anni avete boicottato - sì, lo avete fatto volutamente - il piano di potenziamento dei centri per l'impiego, per i quali avevamo messo in campo, durante il Governo Conte I, un miliardo di euro, con lo scopo di assumere 11.600 nuove unità di personale. Sapete quante persone sono state assunte alla fine del 2022? Appena 4.000: complimenti, avete fatto un ottimo lavoro. Ma alla maggioranza e al Governo di tutto questo non interessa niente; anzi, creare cittadini di serie A e cittadini di serie B sembra un preciso obiettivo e i cittadini di serie B si sentono dire da tempo che, se non trovano lavoro, la colpa è loro. loro. Vi prego, basta con gli *slogan* come il blocco navale, miseramente infrantosi contro i numeri quintuplicati degli sbarchi e l'incapacità di ottenere risposte vere in Europa. Basta con le promesse non mantenute, come quelle sulle accise sui carburanti, che dovevate cancellare, mentre sappiamo bene che avete cancellato gli sconti che le avevano limitate. Basta ancora, vi prego, prego, con gli attacchi alle misure del MoVimento 5 Stelle, con cui pensate di colpire noi come avversari politici e, invece, non fate altro che giocare sulla pelle di lavoratori e famiglie. Basta distrazioni di massa, parlando di sostituzione etnica o di maternità surrogata per nascondere i diritti che nel frattempo calpestate. Pensate veramente di sfasciare l'Italia senza che nessuno se ne accorga? E non parlo di noi qui in Aula, no. Parlo dei cittadini, che inevitabilmente vedranno cadere, una ad una, tutte le vostre maschere classiste e ipocrite. Noi saremo qui a denunciare ogni giorno le vostre azioni ingiuste e sbagliate. Il MoVimento 5 Stelle non arretrerà di un millimetro nel presidiare e difendere quelle idee di Stato solidale e di giustizia sociale che sono alla base della nostra Costituzione. Concludo, Presidente, perché noi vogliamo comunque proporre e costruire. Pertanto rinnovo due proposte concrete che potreste, anzi dovreste cogliere al volo, per dare risposte vere a chi è in difficoltà: salario minimo, per cancellare la vergogna di contratti di lavoro sotto la soglia di povertà da contratti collettivi nazionali e decontribuzione per gli aumenti dei salari, quando la coperta troppo corta del taglio del cuneo fiscale a dicembre esaurirà i suoi effetti. Vi prego: smettetela una volta per tutte di girarvi dall'altra parte. *(Applausi)*.

Signor Presidente, colleghi, Governo, prima di iniziare questo breve intervento vorrei ringraziare il Presidente e tutti i componenti della Commissione, soprattutto la nostra relatrice, per l'ottimo lavoro svolto al fine migliorare il provvedimento oggi in discussione, destinato a cambiare - a differenza di quanto ho sentito dire proprio ora - le sorti dell'Italia e degli italiani, la cui vita dipende dal lavoro. E mi riferisco non soltanto al tipo di vita che ciascuno può condurre in base a quanto può spendere, ma anche e soprattutto alla realizzazione individuale e alla dignità che il lavoro garantisce, migliorando la persona e di conseguenza la società. Non per nulla la Costituzione si apre con l'articolo 1, ponendo il lavoro come base fondante della nostra Repubblica; fondamento però che, a dispetto dei tanti proclami

di quei diritti e di quelle misure che hanno massacrato il lavoro, irrigidendo e soffocando il mercato del lavoro, tartassando datori e lavoratori di tasse, frenando gli investimenti e la crescita, aiutando però la finanza, ma mai le persone, le imprese, le famiglie e i cittadini, cioè il mondo reale. Ci troviamo quindi oggi a dover porre rimedio ai disastri fin qui compiuti e lo facciamo proprio ripartendo da quel mondo, dalle persone, dalle loro necessità, dalle imprese che fanno girare l'economia, creando benessere, con con provvedimenti che ridanno finalmente fiato al mercato del lavoro e garantiscono nuove vie di ingresso per chi può lavorare, prevedendo parallelamente adeguati mezzi di sostentamento e di inclusione per chi non può; inclusione che però non è assistenzialismo strumentale - come è stato finora - ma assistenza mirata a parificare le opportunità e a garantire una partecipazione attiva alla vita della società. Riguardo al reddito di cittadinanza, voglio solo partire da un dato: 18,8 per cento. Che cos'è? È il numero in percentuale dei precettori del reddito di cittadinanza che, secondo ANPAL, a fine 2022 avevano un'occupazione; meno di una persona su cinque, peraltro con impieghi trovati per lo più non grazie al meccanismo del reddito, ma per altre vie. Basterebbe solo questo dato, a distanza di tre anni, per dimostrare e certificare il totale fallimento di questa misura tanto cara ai 5 Stelle. Ma vado oltre. Degli oltre 725.000 percettori del reddito tenuti a sottoscrivere il patto per il lavoro, solo il 42 per cento, cioè meno della metà, si è presentato ai centri per l'impiego per avviare l'*iter* di ricerca di un impiego; percentuale che si abbassa ulteriormente al Sud, dove invece il numero dei beneficiari è sensibilmente maggiore e c'è più bisogno di trovare lavoro. Anche questo dimostra come il reddito abbia totalmente fallito. Queste 725.000 persone occupabili hanno continuato a percepire il reddito di cittadinanza senza essersi mai attivate per trovare un impiego. Fra l'altro, vorrei sapere che fine hanno fatto i navigator, persone la misura è stata sempre un semplice contributo assistenzialistico senza benefici in termini di investimenti, né su se stessi né per la società. Esse non sono state inoltre accompagnate verso un percorso lavorativo. Tale misura non ha agito da moltiplicatore per l'economia, ma ha semplicemente rappresentato una spesa, un esborso improduttivo di denaro pubblico che lo Stato oggi non può e non deve permettersi. Voglio anche citare un altro dato: il 71 per cento dei beneficiari del reddito di cittadinanza ha al massimo il titolo di scuola media. quindi persone non appetibili per le imprese; sono persone che vanno riqualificate. Si tratta di un esercito di potenziali *poor workers*, lavoratori poveri, che non sono in grado di emanciparsi dalla povertà né di aiutare l'economia. Partendo da questi dati, non possiamo che concludere che il reddito di cittadinanza ha avuto solo effetti negativi, a partire da una gravissima deresponsabilizzazione anche morale. È infatti veramente scioccante che oltre la metà dei beneficiari abbia meno di quaranta anni. Che dignità ha uno Stato - chiedo - che invece di porre le condizioni per creare posti di lavoro e garantire l'occupazione dei suoi figli, si limita a offrire loro solo sostegni? Che generazione di cittadini stiamo plasmando? Una platea di futuri adulti incapaci di di provvedere a se stessi, a fronte di migliaia di offerte di lavoro che restano senza risposta, con centinaia di aziende che non trovano manodopera; giovani che sono stati abituati da voi ad avere le loro piccole entrate senza darsi da fare; una stortura terribile voluta da chi ora dalle piazze grida e invita a mascherarsi, con il PD il passamontagna per fare le brigate di cittadinanza. Sono parole irresponsabili e gravissime che non avreste dovuto nemmeno pensare di dover pronunciare *(Applausi)*, soprattutto in uno Stato come il nostro che ha vissuto gli anni di piombo. Vergognatevi quindi e chiedete scusa ai vostri giovani e ai cittadini per lo stato di precarietà in cui li avete ridotti, anche per il ruolo che loro stessi vi hanno affidato e che voi avete offeso e tradito adesso e con il reddito di cittadinanza che è servito solo a pulirvi la vostra coscienza, come se dare un contentino al popolo sia il modo giusto in cui declinare la propria missione di suo rappresentante. No, questo non è il modo giusto. Questo è il solo modo con cui garantirsi consenso al momento debito, facendo leva sul bisogno con cui legare al doppio filo doppio filo chi riceve il debito, esattamente come avviene nei territori di mafia. È una strategia che peraltro non vi è riuscita se oggi sedete nei banchi dell'opposizione. A dispetto di quanto ha affermato il vostro *leader* in piazza l'altro giorno, questa è la piazza della maggioranza del Paese che vede il Governo che non ha soluzioni; 20.000 persone in quella piazza non penso che rappresentino una maggioranza del Paese, ma sono solo le poche rimaste a sostenere le vostre politiche e quelle del PD, della segretaria Schlein che ha voluto affiancarvi e che ogni giorno crea attorno a sé il vuoto. vuoto. Voi avete costruito solo un popolo di precari ed emarginati. Noi oggi cerchiamo di ricominciare a costruire persone, dignità e lavoro. Su questo decreto-legge, come su tutti gli altri ovviamente, ci avete sempre attaccato, additandoci ancora una volta come disumani e disattenti verso le fasce deboli. Ecco questa è una menzogna macroscopica che i fatti smentiscono, partendo anzitutto dall'assegno di inclusione che introduciamo come assistenza alle persone disagiate e bisognose. Parlo di assistenza e non di assistenzialismo, perché prevediamo incentivi per i datori di lavoro incentivi per i datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'assegno e altresì incentivi per l'occupazione giovanile. Prevediamo un beneficio aggiuntivo di sei mensilità dell'assegno per i beneficiari che avviino un'attività autonoma di lavoro, un'impresa o una società cooperativa; il fondo di 7 milioni di euro per gli enti del terzo settore che assumono persone con disabilità. Rifinanziamo i CAF, che normalmente sono di aiuto alle persone meno abbienti; maggioriamo l'assegno unico universale; detassiamo per una quota più alta, e cioè fino a 3.000 euro, i premi aziendali e i rimborsi per bollette per chi ha figli; proroghiamo il *bonus* trasporti; istituiamo l'osservatorio per la povertà. Riduciamo il cuneo fiscale fra il 6 e il 7 per cento per i redditi fino a 35.000, consentendo un aumento sensibile nelle buste paga che dà anch'esso fiato ai lavoratori: misura che avete, anche questa, criticato perché non è strutturale, ma mi chiedo voi cosa avete fatto in questi anni. Queste sono, per grandi linee, le misure che riguardano le fasce più deboli, più povere e più disagiate e i minori, anche aiutando le famiglie

A proposito, a chi in Commissione addirittura piangeva all'idea che a un percettore occupabile si sia offerto un lavoro lontano da casa, voglio dire che dimentica - ed è anche offensivo - che noi dal Sud siamo costretti a emigrare per lavorare da oltre un secolo e che noi mamme del Sud vediamo ogni giorno i nostri figli lasciare la famiglia, gli amici, il lavoro, la propria terra e lì sì che piangiamo, ma non li fermiamo perché non ne abbiamo il diritto se l'opportunità di formarsi, lavorare e realizzarsi è altrove. Piuttosto, quello che stiamo cercando di fare è cambiare questa realtà e dovreste impegnarvi anche voi per farlo, anziché piangere lacrime di coccodrillo per non essere riusciti a costruire il futuro dei nostri ragazzi e avere invece solo distribuito assegni

il potenziamento dell'istruzione, i nuovi contratti collettivi, i finanziamenti per la disabilità, lo sblocco degli appalti e delle grandi opere, la politica del Sud.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, per questo decreto-legge è stata scelta la parola lavoro, una parola che porta con sé un concetto sacro, sinonimo di dignità. Per quanto ci riguarda - e approfitto di questo momento per ringraziare le colleghe e i colleghi con cui abbiamo lavorato in Commissione nelle ultime settimane - questo decreto non è all'altezza di un concetto così sacro e importante. Avevamo provato a inserire alcune proposte emendative, ma purtroppo abbiamo registrato un atteggiamento di netta chiusura; una chiusura che ha significato ad esempio la bocciatura del nostro emendamento che voleva ripristinare la natura universalistica del reddito di cittadinanza, perché si è poveri a seconda non dell'età, ma delle condizioni economiche e sociali e questo - a nostro avviso - è inconcepibile. Vi siate convinti che i percettori di reddito siano tutti dei fannulloni - questo avete raccontato al Paese

Lo sapevamo sin dall'inizio: ci distingue una netta diversità di visione del mondo e del mercato del lavoro. Per voi la competitività delle imprese si incentiva comprimendo e sacrificando sempre e solo i salari dei lavoratori. Per noi non ci può essere incentivo che non tenga conto anche della crescita salariale dei lavoratori. Questa visione, peraltro, è anacronistica, non ha mai funzionato e non la chiedono neanche le imprese virtuose, che sono la stragrande maggioranza in questo Paese, che semmai hanno bisogno e chiedono di investire di più sul capitale umano. Aggiungo che quello dei salari è un tema su cui servirebbe un investimento forte in un momento di forte inflazione, in cui i tassi logorano il potere d'acquisto dei lavoratori e famiglie, ma dal Governo non arriva alcuna risposta. Al contrario, ancora una volta assistiamo alla precarizzazione del mercato del lavoro. Ritornano i *voucher* e non c'è un investimento serio su contratti stabili e di qualità. È stato detto che siamo contrari al taglio del cuneo fiscale: niente di più falso. Voglio ricordare che lo abbiamo fatto per primi, come Partito Democratico. Semmai è vero il contrario, e cioè che con i nostri emendamenti abbiamo provato a rendere strutturale il taglio che voi avete previsto fino al 31 dicembre, anche qui restando totalmente inascoltati. Oltretutto, per fare questo taglio avete trovato le risorse necessarie proprio dallo smantellamento del reddito di cittadinanza (circa 3,5 miliardi di risparmio), alimentando così una guerra tra più poveri e un po' meno poveri. Lo dico con profondo rammarico e pensando anche alla grande attenzione che questo Governo dice di voler avere sul tema della denatalità: pensare di combatterla, creando un mercato del lavoro così come lo state immaginando e costruendo, a me sembra sia in controtendenza rispetto agli obiettivi sbandierati in campagna elettorale e che continuate a sbandierare. Vedete: quando si parla di povertà e di fragilità, a me appare sempre molto normale che la discussione e il dibattito politico e parlamentare si accendano. Il contrasto alla povertà e la rimozione delle ingiustizie e delle fragilità sono spesso alla base del nostro impegno politico. Ho iniziato a far politica occupandomi del mio quartiere e poi della mia città, come consigliera comunale a Pisa. Quando si è trattato di andare al governo della mia città, non ho esitato un secondo a chiedere la delega alle case popolari. Una casa popolare aveva dato alla mia famiglia la possibilità di vivere sotto un tetto e con dignità e a me, nello specifico, di crescere e studiare. Ecco perché, quando si parla di queste tematiche, sento un particolare coinvolgimento, innanzitutto umano. umano. Sono convinta che il Governo e la maggioranza che lo sostiene abbiano ben presenti le difficoltà che vivono tanti nostri concittadini. Mi sorprende pertanto che la risposta a queste difficoltà si concretizzi nella distruzione di una misura di sostegno alla povertà come il reddito di cittadinanza, che presenta due caratteristiche fondamentali: è universale e strutturale. Sono due caratteristiche che accomunano tutte le misure di contrasto alla povertà presenti negli ordinamenti dei Paesi europei. L'Italia, sotto questo aspetto, si era adeguata agli standard europei con colpevole ritardo, e adesso torniamo ancora una volta indietro. Certo, a distanza di qualche anno dalla sua introduzione, il reddito di cittadinanza poteva essere migliorato, ma una cosa è certa: questo provvedimento aveva rappresentato per l'Italia un grande passo avanti sul tema del contrasto alla povertà che, a discapito del nome, ha svolto il ruolo di reddito minimo garantito, così come lo conosciamo in altri Paesi europei. Questo lo diciamo non noi, ma i numeri: tale misura, soprattutto in una fase di grande difficoltà come quella che abbiamo vissuto in occasione della pandemia, ha dato sostegno a migliaia di famiglie. Ciò che serviva era migliorare e potenziare la presa in carico del percettore di reddito in un percorso di ricollocamento o di inserimento nel mercato del lavoro. Su questo aspetto avremmo potuto lavorare insieme per ovviare ai problemi e ai limiti che sono emersi, ma avete deciso di fare in altro modo. Per tutti i poveri occupabili poi viene anche rafforzato l'obbligo di accettare qualsiasi lavoro che garantisca i minimi contrattuali, a prescindere dai costi di trasporto ed eventuale soggiorno, insomma senza tenere conto della congruità dell'offerta di lavoro. Su questo punto in seguito le mie colleghe. Certo, è positiva l'attribuzione ai servizi sociali comunali della valutazione multidimensionale della situazione della famiglia e dei singoli componenti. L'unica pecca è che non c'è un solo euro permettere ai Comuni di svolgere questo compito nel miglior modo possibile. Infine, avviandomi alla conclusione, non si comprende in quale modo e con quale stratagemma le politiche attive del lavoro, che sono state il pezzo mancante delle riforme finora attuate, dovrebbero e potrebbero funzionare. Era lì lì che bisognava intervenire, ma di questo, che era davvero il punto più importante da rivedere e da far funzionare, il decreto-legge non si occupa. È chiara la gravità del fatto che, con il provvedimento in discussione, l'Italia non solo non fa alcun passo avanti sul tema della povertà e del lavoro, ma anzi ne fa più di qualcuno indietro. Avevamo una grande occasione: recuperare il *gap* sulle politiche attive del lavoro e migliorare le inefficienze sulle misure di reddito minimo. Avete deciso di non fare né l'una né l'altra cosa. Avete deciso di alimentare una guerra tra poveri e meno poveri: ne pagheranno le conseguenze tante famiglie italiane e tanti cittadini che si sentiranno nuovamente abbandonati dallo Stato. *(Applausi)*.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, l'Assemblea del Senato si trova in questa giornata a discutere un testo davvero importante, che incardina misure volte ad incidere su due temi fondamentali per la nostra società:

non una scelta casuale, non una scelta di facciata, ma una scelta di merito, perché introduce, in un contesto e in una giornata significativa, misure importanti a tutela del lavoro e dei lavoratori. L'obiettivo è, infatti, quello di aumentare stabilmente l'occupazione, tagliare il cuneo fiscale e attuare misure per abbassare gli effetti dell'inflazione sulle buste paga degli italiani. Dopo i massicci interventi per contrastare il caro bollette inseriti nella legge di bilancio, che hanno consentito di abbattere i costi di luce e gas, l'attenzione del Governo si è concentrata sull'obiettivo di aumentare il potere di acquisto delle famiglie italiane. Stiamo intervenendo con misure concrete ed efficaci rispetto ai tanti e gravi problemi che ci avete lasciato e che pesano sulla vita quotidiana degli italiani, soprattutto dei più deboli. Il decreto-legge introduce una serie di provvedimenti a sostegno dei lavoratori, dell'occupazione, ma anche delle imprese, il più importante dei quali è certamente quello relativo al taglio delle tasse sul lavoro.

Sono state liberate risorse per circa 4 miliardi di euro, che il Governo ha voluto destinare al taglio del cuneo contributivo di quattro punti percentuali, che si vanno a sommare al taglio che già era stato introdotto con le misure contenute nella legge di bilancio. Ciò consente di realizzare ora un taglio del cuneo contributivo di sei punti percentuali per i redditi fino a 35.000 euro e di sette punti percentuali per i redditi più bassi, quelli fino a 25.000 euro. In un periodo in cui crescono sia il costo della vita che l'inflazione,

sta dimostrando di saper mettere da subito concretamente in atto, in assoluta coerenza con il mandato ricevuto dagli italiani. L'attenzione alle famiglie e ai più fragili si conferma anche con altre misure, come l'incremento a 3.000 della soglia dei *fringe benefit* aziendali per i lavoratori con figli a carico. Questi sono aiuti concreti, perché sono buoni spesa o buoni pasto che saranno interamente detassati. Si prevede, inoltre, un'estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell'assegno unico per i figli: misure concrete, che vanno a incidere su quello che è il nucleo fondamentale della nostra società, la famiglia, attorno alla quale tutte le politiche del Governo Meloni si stanno muovendo con azioni concrete ed incisive. Per contrastare la povertà e l'esclusione sociale, con particolare attenzione alle famiglie al cui interno siano presenti soggetti fragili, minori o anziani, dal 1° gennaio 2024 verrà attivato l'assegno di inclusione. Il beneficio mensile, che avrà un importo non inferiore ai 480 euro, verrà erogato dall'INPS quale integrazione al reddito, in favore di quei nuclei familiari che comprendono appunto persone con disabilità, minori e ultrasessantenni che siano in possesso di determinati requisiti; avrà una durata di diciotto mesi e potrà essere rinnovato per altri Per attivare questo beneficio i destinatari dovranno sottoscrivere un patto di attivazione digitale che preveda anche incontri trimestrali per l'aggiornamento della propria posizione. Noi abbiamo sempre sostenuto che non è corretto che uno Stato metta sullo stesso piano chi non può lavorare e chi invece può farlo. Per questo confermiamo, e anzi oggi miglioriamo il sostegno per chi non può lavorare: famiglie in difficoltà, nel cui nucleo ci siano persone con disabilità, minori, bambini o anziani. Chi può lavorare viene invece inserito in un percorso di formazione o riqualificazione al lavoro, prevedendo però di garantirgli un rimborso spese pari a 350 euro nel periodo in cui avviene questa formazione e prevedendo altresì incentivi importanti per chi dovesse assumere chi è entrato in questo percorso. È un cambio di paradigma rispetto al reddito di cittadinanza, in cui venivano invece diseducati alla ricerca del lavoro e in cui - possiamo dirlo - i dati sono stati chiari, anche nelle numerose audizioni che abbiamo avuto: questa misura ha completamente fallito per quanto riguarda la sua vocazione di politica attiva del lavoro. Si è trasformata in una misura assistenziale, disincentivando di fatto la ricerca del lavoro, che è invece una pietra miliare non solo della nostra Costituzione, ma anche di quel valore, di quella dignità che il lavoro porta con sé per tutti i cittadini italiani. Abbiamo talmente a cuore i nostri giovani, a differenza di quello che ho sentito dire e che si è scritto in questi mesi e nelle ultime settimane, che vogliamo investire realmente su di loro. Per questo, per incentivare l'occupazione giovanile, sono previsti incentivi pari al 60 per cento delle retribuzioni, a favore di quei datori di lavoro che assumono giovani di età inferiore ai trent'anni. Questo decreto si occupa anche del lavoro delle persone con disabilità, sostenendone l'assunzione da parte degli enti del terzo settore, con appositi incentivi e il relativo fondo di finanziamento. Con le misure previste si interviene anche per il rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni e con specifici controlli ispettivi. Siamo stati tutti drammaticamente colpiti dalla mole di infortuni, anche mortali, che hanno coinvolto ragazzi impegnati nell'alternanza scuola-lavoro. Per questo si è intervenuti con una revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative. Sempre in tema di sicurezza sul lavoro, sono previsti, ad esempio, l'obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente, se richiesto dalla valutazione dei rischi; l'estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; l'obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di particolari attrezzature e attività attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza. In conclusione, Presidente, le misure che andremo ad approvare oggi hanno visto un approfondito *iter* in Commissione, che ci ha visti udire e confrontarci fattivamente con moltissimi soggetti. Per questo mi sento di ringraziare *in primis* la senatrice Mancini per il grande lavoro svolto, il Presidente e tutti i membri della Commissione. Noi guardiamo con attenzione al mondo del lavoro, con questo atto in approvazione, taglio del cuneo fiscale; gli incentivi alle assunzioni; la presa in carico dei soggetti più fragili; la formazione retribuita per aiutare chi può ad entrare nel mondo del lavoro; interventi sulla sicurezza; gli incentivi per l'occupazione delle persone con disabilità, dei giovani, delle donne vittime di violenza; il finanziamento dei centri estivi per conciliare famiglia e lavoro. Sono tutte misure di buonsenso, necessarie e a favore degli italiani, che sono la nostra priorità.

Non è vero che il Governo o la maggioranza sono stati sordi, ma è stato fatto quello che poteva essere fatto, avendo chiara la direzione che si voleva imprimere. infatti una visione strategica, che chiaramente è diametralmente opposta a quella di chi ci ha preceduto al Governo fino ad ora. Negli ultimi anni, chiunque sia in buona fede ha potuto rendersi conto dei danni profondi, spesso difficilmente rimediabili, provocati da scelte politiche dettate non solo da impostazioni ideologiche, ma persino da un puntiglio o da una mossa di mera e sterile propaganda: quella che abbiamo ascoltato anche adesso negli interventi dell'opposizione.

che si accorge degli errori compiuti in precedenza, ha il dovere di affrontare la situazione per quello che è, ponendo rimedio agli errori e ai paradossi, che sono rimasti come un macigno sul percorso dello sviluppo della Nazione. È questo il caso del reddito di cittadinanza. Il fallimento conclamato di una delle battaglie simbolo del MoVimento 5 Stelle si riassume tutto nei dati che arrivano dall'INPS e dall'ISTAT: due terzi dei 3,7 milioni di beneficiari dalla misura, cifra che nel bilancio pubblico impatta per 8 miliardi di euro, pari quindi a 2,4 milioni di individui, non risulta presente neanche negli archivi INPS degli estratti conto contributivi degli anni 2018 e 2019. Tradotto, questo significa che due percettori su tre non solo non hanno trovato lavoro nel periodo di erogazione del reddito, ma proprio non lo hanno cercato. anche si volesse escludere il tema del lavoro dal bilancio del reddito di cittadinanza, le cose non andrebbero meglio. L'ISTAT rivela, infatti, che nel 2020 le famiglie in condizione di povertà assoluta, cioè non in grado di acquistare un paniere di beni e servizi sufficiente a uno *standard* di vita minimamente accettabile, sono aumentate da 1.674.000 a 2 milioni, il che equivale a centinaia di migliaia di Se il reddito di cittadinanza, da una parte, ha permesso a una fetta di popolazione di uscire da un livello di povertà assoluta e probabilmente anche di affrontare il momento apicale della pandemia; dall'altro ha creato nuovi poveri, alterando la geografia della distribuzione dei meno abbienti dal Sud al Nord. Il reddito di cittadinanza può probabilmente definirsi il fallimento per eccellenza, proprio perché contiene in sé l'illusione del successo a buon mercato, ma si è rivelato una misura ben lontana dagli obiettivi per cui era stata progettata. Se poi si riconoscesse che si tratta di uno strumento di assistenzialismo come un altro, si potrebbe anche chiudere qui ogni valutazione. È giunto quindi il momento di acquisire una concezione diversa dello stato di cittadinanza, nel senso di individuare e implementare quelle attività inclusive che trasformano una persona in un cittadino, capace di fare la sua parte in una comunità organizzata, attraverso la dignità del lavoro. Ai beneficiari del reddito di cittadinanza, così come era stato concepito, prima che il lavoro, manca la capacità di divenire un lavoratore. Solo superando questo, si possono diradare le nebbie degli equivoci insiti nel reddito cittadinanza. Il reddito, per stessa ammissione di chi lo ha immaginato, non ha creato occupazione, ma ha svolto un diverso ruolo sociale, che oggi però l'Italia non può più sostenere, né dimensionalmente, né eticamente. Se, da una parte, il sostegno agli indigenti deve continuare e continuerà a essere una priorità sociale del nuovo Governo, non si possono più depauperare le risorse dello Stato che non qualificano il capitale umano, non solo sotto il profilo delle competenze, ma anche da un punto di vista culturale. Il vero danno è la mancata affermazione del valore del lavoro come strumento e mezzo di riscatto e di emancipazione sociale, regalando ai nostri figli l'ennesimo alibi del lavoro che non si trova. In Italia milioni di ragazzi tra i quindici e i ventiquattro anni hanno scelto di non studiare e neppure provano a cercare un lavoro. L'emigrazione dei cervelli, la crisi economica e oggi il reddito di cittadinanza sono diventati un ulteriore alibi per continuare a illudere i nostri figli, destinandoli così alla paralisi e all'emarginazione. È quindi necessaria una scelta molto più difficile di quella che si è limitata - com'è avvenuto in generale fino a ora - a erogare un assegno e a passare oltre, ma è la sola utile a fare avanzare la nostra società. Ed è la scelta di questo Governo, che sta mettendo giù tanti piccoli tasselli per far ripartire il mercato del lavoro. Questa è l'impostazione culturale e politica che è alla base del decreto. Tra le principali novità che voglio sottolineare vi è sicuramente l'istituzione dell'assegno di inclusione, come nuovo strumento che andrà a sostituire il reddito di cittadinanza e che potrà essere richiesto dai nuclei familiari con disabili, minorenni e *over* 60 in possesso di determinati requisiti relativi alla cittadinanza o all'autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche. In sede di esame in Commissione - ambito nel quale, come ho detto prima, è stato svolto un lavoro ampio e approfondito - sono stati apportati importanti miglioramenti, frutto del confronto politico, anche con le tante categorie. In particolare, mi preme sottolineare l'approvazione di un emendamento che ha esteso il riconoscimento dell'assegno ai componenti del nucleo familiare svantaggiati e inseriti in programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione, quale doverosa misura di inclusione da destinare, ad esempio, ai senza fissa dimora e ai minori che fuoriescono dal circuito delle case famiglia per il passaggio alla maggiore grazie all'approvazione un altro emendamento, l'assegno di inclusione potrà svolgere un ruolo fondamentale nel recupero dell'autonomia economica delle donne che hanno subìto violenza, supportandole soprattutto nella prima fase del loro percorso. La possibilità di accedere a un sussidio economico che garantisca una sicurezza economica nel breve e medio periodo, infatti, incide sia sulla scelta della donna di lasciare il maltrattante in caso di convivenza, sia su quella di uscire dalle case di accoglienza. Ha quindi un duplice impatto positivo, permettendo di allontanarsi dalla situazione di violenza e di prevenire eventuali recidive, contribuendo nel contempo a liberare più velocemente le disponibilità di posti dalle case di rifugio, così da consentire a un numero maggiore di donne di essere accolte. Chi ha accusato il Governo Meloni di non occuparsi delle difficoltà delle famiglie italiane dovute al caro vita ha avuto da noi una risposta precisa. Un'altra misura fondamentale e qualificante inserita all'interno del decreto prevede, per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, un 31 dicembre 2023, un importante taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, grazie a un esonero parziale dei contributi previdenziali a loro carico, che potrà portare ad avere fino a 100 euro in più nella busta paga mensile. Inoltre, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, sono previsti dei *bonus* per le assunzioni a favore delle aziende che andranno ad assumere *under* 30 dal 1° giugno al 31 dicembre. Per poter beneficiare dell'incentivo i giovani lavoratori devono avere meno di trent'anni di età, essere Neet, cioè essere persone che non lavorano, né sono inserite in corsi di studio o di formazione, così da poter essere registrati al Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani. Concludo, signor Presidente, dicendo che chiaramente ancora una volta,

con questo decreto noi stiamo definendo un percorso che darà senso alla possibilità di sviluppo economico attraverso il lavoro e non attraverso l'assistenzialismo.

di maggioranza. Devo dire che il rilievo che ha avuto la discussione in Commissione - ringrazio tutti i commissari presenti, di maggioranza e di opposizione - è stato molto alto. Ognuno ha parlato

È vero anche, Presidente, che nella discussione e nel dibattito politico che, dal 1° maggio a oggi, ci hanno accompagnato, sono stati toccati pochissimi temi tra tutti quelli che invece il cosiddetto decreto lavoro tocca. Questo spiace, perché ce ne sono molti di interesse. Ma, chiaramente, soprattutto l'opposizione ha voluto porre l'accento là dove legittimamente, ma incomprensibilmente, è stata fatta solo polemica. Ancora oggi ne abbiamo sentito in quest'Aula, soprattutto da parte di un Gruppo politico, Presidente, che non si rassegna a dover rimettere in frigo le bottiglie vuote di quando si è brindato alla fine della povertà povertà che non è mai finita, ma anzi è aumentata negli ultimi cinque anni. A chi ci dice che il reddito di cittadinanza non doveva essere eliminato - come non lo è stato ma doveva essere modificato e migliorato, rispondiamo che ciò è stato fatto, negli ultimi mesi e in questo decreto, e gli effetti positivi delle modifiche si sono subito visti.

provvedimenti precedenti. In questo in parte gli posso dare ragione: sono merito del reddito di cittadinanza che è stato modificato in positivo. Da quel momento le assunzioni sono schizzate in alto e hanno raggiunto le 500.000 unità: merito del momento positivo trasmesso a chi deve assumere, ma merito anche di tutti quei percettori che, sapendo di non poterla più far franca non poterla più far franca e sapendo che non avrebbero più avuto diritto al reddito, hanno incominciato a cercare e a trovare lavoro. Anzi, a cercarlo non tanto, perché il lavoro era già lì, era solo da cogliere. E così in pochi mesi le assunzioni sono cresciute tantissimo.

che le Regioni, soprattutto quelle del centrodestra - ma poi, vedendo i dati, si equivalgono tutte - hanno boicottato gli elementi cosiddetti positivi del reddito di cittadinanza, a partire dal potenziamento umano e infrastrutturale dei redditi di cittadinanza, raccontate o fate suonare un disco rotto, che si inceppa. Personalmente ho fatto l'assessore al lavoro di Regione Liguria per sette anni e mi sono occupato del potenziamento dei centri per l'impiego. Vi dico che la Liguria, con un'amministrazione di centrodestra e con l'assessore al lavoro di Fratelli d'Italia - pensate voi: il massimo della negatività che voi possiate, è stata la prima a finire il potenziamento in termini di assunzione di donne e uomini nei centri per l'impiego ed è stata la prima a iniziare il potenziamento dei centri per l'impiego dal punto di vista infrastrutturale. *(Applausi)*. E allora cosa raccontate?

Non siamo però allo stadio, ma nell'Aula del Senato, e io naturalmente gliene sono molto grata. Prego, continui, e le verrà conteggiato il tempo tranquillamente. È inutile quindi continuare a raccontare una favola che non c'è. Laddove non si è riusciti a potenziare, le cause vanno cercate in altri fattori e non certo nella volontà politica di affossare un provvedimento che si è affossato da solo.

Così è stato, perché chi era al Governo nella precedente legislatura non ha avuto il coraggio e non ha potuto dal punto di vista legislativo trasformare i contratti co.co.co in contratti a tempo indeterminato. Sapete cosa ha fatto, Presidente? Forse lo sa benissimo e lo sanno anche coloro a cui mi rivolgo tramite lei. hanno scaricati sulle spalle delle Regioni *(Applausi)*, che non hanno potuto fare altro che lasciarli a casa, senza alcuna risorsa in più per poterli stabilizzare. Se non ci riesce il Governo, sicuramente non ci possono riuscire le Regioni. Quando però noi dicevamo queste cose, ci davano dei portatori di iella perché si trattava non di un altolà a chi voleva fare quel provvedimento all'epoca, ma di un tentativo per affossare il reddito di cittadinanza che poi - come sappiamo - si è poi affossato da solo nei risultati. Devo anche dire, Presidente, che

alle storie vere - e ce ne sono tantissime - raccontate in piazza dal MoVimento 5 Stelle. Forse non c'entra con questa discussione, ma vorrei ricordare che, se quelle storie raccontate non fossero state sopraffatte nell'interesse da chi, parlando di lavoro e di dignità, invoca le brigate di cittadinanza e il passamontagna, forse avrebbero trovato molto più interesse anche in questa maggioranza e nei giornali. Non è allora colpa nostra questa disattenzione.

volontà dei datori di lavoro di non dare certezza a chi cerca lavoro, anche solo per un *weekend* o tutti i *weekend* dell'estate. Il superamento del decreto dignità di utilizzare i lavoratori a chiamata e i lavoratori a tempo determinato in determinati settori aiuta e sta aiutando l'economia italiana a superare e lasciarsi alle spalle le crisi che abbiamo passato, e aiuta tantissimi lavoratrici e lavoratori, che cercano lavoro a tempo determinato o che si affidano al lavoro determinato perché altri non ne possono trovare, ad ottenere un lavoro retribuito e protetto dalle assicurazioni e non, come successo negli ultimi anni, a trovare solo lavoro in nero. Un ultimo accenno lo devo fare a chi negli anni del Governo precedente a questo se ne è infischiato di rinnovare i contratti collettivi in aumento, lasciando che continuassero a rinnovare i contratti collettivi senza aumento, per poi dire adesso che noi dobbiamo fare quello che non è stato fatto in alcuno degli ultimi dieci anni da alcuno degli ultimi Governi. Oggi chi è stato al Governo per dieci anni ci dice che gli stipendi per colpa dei contratti collettivi nazionali sono troppo bassi.

oggi siamo chiamati a discutere una proposta di legge che nasce con l'intenzione di offrire risposte alla questione della povertà, al suo dramma, all'inclusione sociale e socio lavorativa. invece a confrontarci su un testo che affronta molte questioni, diverse tra di loro, anche troppo, offrendo però risposte del tutto inadeguate. Sappiamo bene come nasce il decreto-legge, ovvero dalla campagna elettorale emersa continuamente sul tema di come abolire il reddito di cittadinanza, una bandiera di contrapposizione politica, quando invece sul tema della povertà dovremmo avere tutti la stessa bandiera, che è quella del riconoscimento della dignità umana della persona e della famiglia, offrendo delle *chance* per uscire dalla povertà. Con questa proposta di legge si supera ogni tentativo di costruire una normativa che metta il nostro Paese accanto alle grandi democrazie europee nel sostegno della povertà, nelle politiche di inclusione. Addirittura si dividono i poveri per categoria e la discriminante della divisione è l'età l'età anagrafica, come se dipendesse solo da quella lo stato di povertà. La sostituzione del reddito di cittadinanza con l'assegno di inclusione diventa una misura categoriale rivolta esclusivamente a un certo tipo di famiglia con minori, anziani, disabili e tutto il resto viene tralasciato. Abbiamo visto tutti le stime: con la nuova legislazione circa il 50 per cento delle famiglie che oggi hanno il reddito di cittadinanza rimane esclusa da questo tipo di copertura e di sostegno. allora, e credo che ognuno di noi se lo chieda: il resto, l'altro 50 per cento che fine fa? Lo abbandoniamo a sé stesso? Non riconosciamo più a questi il diritto all'inclusione, alla propria dignità? poi la questione dei figli, che è eclatante: a diciotto anni non si è più considerati una parte della famiglia che deve essere sostenuta. sostenuta. Ebbene, in questo Paese la scuola e la formazione, negli anni passati, nel nostro Dopoguerra, ha davvero definito e creato

Abbiamo ascoltato in Commissione tante associazione laiche e cattoliche, fra cui la Caritas, che ogni giorno è in campo contro la povertà, e tutte ci hanno detto una cosa: non va bene non riconoscere la povertà per tutti quelli che hanno questa condizione. L'occupabilità della persona non è soltanto un dato anagrafico, ci sono tanti fattori, anche quello formativo, anche quello culturale, anche quello del disagio sociale, anche quello delle dipendenze, che la determinano. Come si fa a discriminare i poveri? Credo che questa sia la cosa più grave che stiamo facendo e siccome quando si tratta della dignità delle persone divento ostinata e testarda,

poi il tema di come si riconosce la possibilità dello sbocco lavorativo. Questo è un tema delicatissimo e importante, perché significa creare davvero per le persone l'uscita dallo stato di povertà. Se c'è una cosa che ha funzionato poco nel reddito di cittadinanza è stata proprio la seconda gamba, l'occupabilità delle persone.

È vero, in alcune Regioni del nostro Paese, tra cui - in modo un po' più parziale rispetto a quello che ho ascoltato - la Liguria,

Qual è l'accompagnamento formativo che deve essere un diritto per chi cerca lavoro e, in modo particolare, per chi cerca lavoro per uscire dalla povertà? Non abbiamo visto alcun investimento

non l'abbiamo più vista: *desaparecido.* Dopo l'annuncio di un confronto importante in Commissione sul progetto delle politiche attive del lavoro, non abbiamo più avuto modo di incontrarla, di discuterne e nemmeno di ascoltare i progetti che si vogliono portare avanti. Inoltre, non si combatte la povertà creando condizioni per una corsa ad ostacoli per chi è povero:

Ma ci si rende conto di cosa stiamo parlando? Quando si tratta del lavoro, che è la vera condizione di dignità della persona, si deve parlare con il grande rispetto che si ha per la coesione sociale, per il valore sociale del lavoro e soprattutto per la dignità umana di qualsiasi persona. Mi soffermo sul tema del lavoro.

Vogliamo ancora allargare questo stato? Quando pensiamo di legare il rinnovo, la cosiddetta deroga, alla possibilità di contrattazione diretta tra l'azienda e il singolo lavoratore precario, pensiamo davvero che ci sia la stessa forza da una parte e dall'altra del tavolo? Io credo di no.

non bastava averli ripristinati: addirittura li allarghiamo, tra l'altro in uno di quei settori che hanno una flessibilità contrattuale direi davvero estrema.

che sia possibile almeno per alcune categorie, a partire ad esempio dai lavoratori fragili, creare le condizioni affinché sia possibile in quest'Aula perché gli strumenti che abbiamo davanti e di cui dobbiamo discutere sono seri e sono legati innanzitutto alla serietà che dobbiamo agli uomini e alle donne del nostro Paese.

si propone di ripristinare il fondo che la ministra Calderone aveva abolito alcuni mesi fa. Questo è ciò che avviene, quindi siamo di fronte al fatto che si ritiene di

di venire a lavorare nel mio Paese non accetta la proposta, perde il diritto. Questo non esiste. Sappiamo tutti che c'è un problema di rapporto tra domanda e offerta, c'è un problema di quali condizioni

avete tolto le causali e avete liberalizzato. Si può arrivare a ventiquattro mesi senza una causale, perché si stipula un contratto a termine; addirittura si introduce il fatto che le causali si possono determinare tra il singolo lavoratore o lavoratrice e il datore di lavoro. Come tutti ben sanno, ben sanno, non c'è parità di condizione quando si contratta in questa situazione: questo è il dato. È un terreno di subalternità e mettete in difficoltà le persone da questo punto di vista. Non ci avete ascoltato assolutamente, su niente.

parliamoci chiaro: sono passati nove mesi da quando siete al Governo. La dovete smettere di continuare a pensare che la colpa è degli altri. Dovete dire che cosa fate voi.

Avete allargato le maglie per i datori di lavoro che chiedevano maggiore flessibilità: questo è il dato. Invece, ovviamente, non avete avanzato non avete avanzato una proposta per cercare di affrontare il problema della perdita del potere d'acquisto dei salari. Per fortuna, in qualche modo, qualche contratto si sta rinnovando. Ieri è stato rinnovato il contratto del legno e affini, il contratto dei meccanici prevede un recupero del 6,6 per cento dell'inflazione; questi rinnovi aumentano la paga base, migliorano le condizioni dei lavoratori e la loro disponibilità economica, perché quando si aumenta la paga base c'è un rapporto con l'insieme

sia considerato come parte della retribuzione, una specie di salario "mordi e fuggi". Davvero pensate di costruire una società in questo modo?

di ridurre la precarietà, di prevedere delle assunzioni programmate, di dare certezza, di mettere in condizioni chi ha studiato di svolgere un ruolo e una funzione per quello che ha appreso durante il suo studio. Questa è la cosa da fare: parlare di lavoro e offrire le occasioni di lavoro. Voi invece pensate di dare solo al mercato la condizione per creare i posti di lavoro. Guardate, io non sono contro l'impresa, so benissimo che se esistono i lavoratori esiste anche un'impresa. Il problema è se l'impresa ha delle regole, oppure è tutto libero, purché - come si usa dire - ci sia un posto di lavoro. Questo non avviene. Discutete di lavoro, ma tutto questo non c'è. Tutto questo, in questo decreto, non c'è. L'unica cosa che c'è in questo decreto è maggiore precarietà e maggiore flessibilità.

al mondo del lavoro e ai lavoratori. Purtroppo, per colpa della maggioranza, è impossibile dare questo contributo e quindi voteremo contro il provvedimento in

Secondo quanto afferma il Governo, lo scopo del provvedimento è quello di agevolare e promuovere la trasparenza e la semplificazione del mondo professionale. che tutti voi possiate essere d'accordo sul fatto che temi così importanti, come la promozione dell'inclusione e la tutela del mercato del lavoro, necessitino di un impianto normativo coerente nel suo insieme, dotato di una visione volta a risolvere non solo le urgenze momentanee, ma anche a garantire una prospettiva di lungo periodo. Un primo punto che vediamo in modo favorevole riguarda certamente l'inserimento dell'assegno di inclusione, che andrà a sostituire, già a gennaio 2024, il reddito di cittadinanza oggettivamente, è un provvedimento che ha disatteso le aspettative, come del resto molti di noi avevano previsto sin dal principio, in tempi non sospetti, quantomeno per come era scritto e applicato. È una scelta che riteniamo eticamente ed economicamente più corretta, che servirà a sostenere quelle persone che dimostrino oggettivamente di non essere in grado di lavorare, cercando di non lasciare nessuno indietro. L'intento è valido e condivisibile, però crediamo che tutte le misure di sostegno al reddito debbano essere eque, effettive ed universali. È proprio con riguardo all'universalità della misura che nutriamo qualche dubbio sulla sua reale applicazione. Ad esempio, devo rilevare la rigida individuazione dei criteri per poter beneficiare dell'assegno di inclusione. Questo, infatti, comporta il rischio di escludere i soggetti senza fissa dimora, per fare un esempio, che in quanto ultimi tra gli ultimi dovrebbero poter fruire di misure di sussistenza, così come già segnalato anche da numerose associazioni di categoria, che sono state audite in Commissione. Un'altra criticità attiene a un ambito a me molto caro: parlo del mondo della disabilità. Riprendendo le perplessità già manifestate anche dalla Federazione italiana che l'attuale formulazione della norma comporta due sostanziali rischi, che non sono assolutamente da sottovalutare. Il primo è che l'assegno di inclusione, così come disciplinato, rischia di escludere persone con disabilità che non rientrino nelle ipotesi di disabilità media, grave o o non autosufficiente. Sarebbe opportuno, decisamente opportuno, estendere la misura anche a quei nuclei familiari che presentano un componente con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3, della legge n. Il secondo aspetto che deve essere chiarito è che, dal calcolo del reddito familiare a cui far riferimento per poter beneficiare dell'assegno di inclusione, devono essere escluse espressamente le prestazioni connesse all'invalidità civile. Riguardo a questo punto, voglio specificare che il testo di questa norma è poco chiaro e consideriamo assolutamente necessario intervenire per evitare che i percettori di assegno di invalidità civile o di pensione di invalidità siano ingiustamente discriminati. Peraltro, parliamo di assegni e di pensioni che si aggirano intorno ai 300 euro: sarebbe pure più dignitoso definirli Come detto, il provvedimento in discussione presenta punti di forza e di debolezza. Chiaramente positiva è la parte che riguarda la riduzione del cuneo fiscale di 4 punti percentuali, per i lavoratori dipendenti con reddito lordo fino a 35.000 euro, assunti per il periodo che va dal 1o luglio al 31 dicembre. Indubbiamente è un passo in avanti, per contrastare il costo della vita e per incentivare i consumi. Occorre però che il costo del lavoro diminuisca ulteriormente, che la misura divenga strutturale e non occasionale o per soli quattro mesi, come in questo caso *(Applausi)*. Serve infatti che sia rifinanziata nella prossima legge di bilancio e per i prossimi anni, prevedendo maggiori riduzioni del costo del lavoro, anche per la quota a carico del datore di lavoro. Se non si interviene seriamente, questo tipo di azioni non può essere considerato buono o idoneo per tanti datori di lavoro, né tantomeno potrà stimolare nuove assunzioni. Voglio ricordare in quest'Aula che proprio l'abbattimento del cuneo fiscale è stato da sempre un cavallo di battaglia del centrodestra, motivo per cui oggi ci aspettiamo più coraggio e più convinzione *(Applausi)*, affinché l'Italia non venga più annoverata come uno dei Paesi OCSE con il peso del cuneo fiscale più alto: alto: voglio ricordare che già oggi supera il 45 per cento. Da condividere è anche la previsione di misure per rafforzare l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che possono certamente prevenire le cosiddette morti bianche, morti inutili e ingiuste su cui bisogna assolutamente intervenire proprio per migliorare la vigilanza e la sicurezza. Altro aspetto che ci inorgoglisce e che voglio ricordare

a me sta particolarmente a cuore, è quello legato agli incentivi per il lavoro delle persone con disabilità. Mi riferisco nello specifico all'articolo 28, che istituisce un fondo di 7 milioni di euro per il 2023, finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e non lucrative che assumono, ai sensi della legge n. 68 del 1999, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tra il 1° agosto del 2022 e il 31 dicembre del 2023, persone con disabilità di età inferiore a trentacinque anni. Ci verrebbe da dire finalmente e vi verrebbe da dirlo insieme a me. me. Guardare alle persone con disabilità non più come un peso, ma come una risorsa per la società, era forse un sogno troppo ambizioso fino a qualche tempo fa. fa. Oggi sembra realtà, ma ci si imbatte nei labirinti dei decreti attuativi, che invece ci riportano alla cruda realtà e dai decreti attuativi dipende praticamente tutto. Il decreto in discussione oggi, infatti, demanda l'individuazione di modalità e procedure a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la disabilità, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro

di concertazione tra Ministri competenti: il nostro invito è che vi concertiate prima *(Applausi)* e, al riguardo, ho pensato di darvi una mano, non per gentilezza, ma per spirito di squadra, per spirito costruttivo, affinché nessuno davvero resti indietro, ma perché si possano offrire risposte serie. Approfitto, quindi, per ricordare a tutti i colleghi presenti e al Governo che tra gli emendamenti che ci apprestiamo a esaminare e a votare ce n'è uno, a mia prima firma, proprio all'articolo 28, con il quale si prevede che il fondo possa vedere la luce non dopo dieci mesi, ma dopo tre, un tempo che mi sembra più che sufficiente, soprattutto se si pensa che l'operazione non comporta oneri di spesa aggiuntivi. Forse tre mesi vi sembrano pochi? Allora riformulatelo per non andare oltre dicembre 2023. Onestamente lasciare la data del 1° marzo 2024 è una vera esagerazione: vorrebbe dire quasi dieci mesi di attesa per un decreto attuativo. Signor Sottosegretario, mi rivolgo a lei per il tramite della Presidenza, perché conosco anche la sua sensibilità. Non ci sono oneri di spesa aggiuntivi. Rivedete il termine per il decreto attuativo. *(Applausi)*. Il mio emendamento, il 28.101, vi dà proprio la possibilità di correggere il tiro e dare risposte rapide e serie anche al mondo del terzo settore, motivo per cui colgo l'occasione di chiedere, anche a tutti i colleghi di maggioranza e opposizione, di soffermarsi sulla Ridimensionare le tempistiche per l'emanazione dei decreti attuativi è urgente e necessario e non lo chiedo solo io, ma milioni di persone e numerose associazioni che hanno più volte sollevato il tema anche nel corso delle audizioni in Commissioni, citarne una tra tutte, Confassociazioni. Certo, un altro punto su cui ci sarebbe piaciuto trovare più spazio e modalità di discussione sarebbe stato il salario minimo. A nostro avviso si tratta di un traguardo di civiltà, ma questo è un altro capitolo. Vado a concludere, Presidente. Mi sento di dire che questo provvedimento sicuramente presenta dei punti interessanti, ma decisamente ancora migliorabili, quindi il mio auspicio è che il Governo abbia la giusta attenzione e sensibilità per valutare seriamente i suggerimenti che abbiamo presentato con lo scopo di migliorare questo testo che a breve ci approcciamo a discutere e a votare.

il decreto-legge contiene in primo luogo nuove misure di inclusione sociale e lavorativa. Cambia cioè l'approccio alla lotta alla povertà e alle situazioni di marginalità. Si tratta di un nuovo modo di includere chi ha più difficoltà, senza quindi lasciare indietro nessuno; oltre a prevederne l'inserimento nel tessuto sociale, si responsabilizza chi percepisce un assegno dello Stato. Questa è la ragione che sostiene l'introduzione dell'assegno di inclusione.

che vedevano la partecipazione nel mondo del lavoro che aveva il reddito di cittadinanza. Al contrario, si pone come obiettivo quello di coniugare la necessità dei sussidi per chi non lavora con la presenza di politiche attive del lavoro che siano efficaci. L'assegno va alle famiglie con minori disabili e torna ad essere un sostegno per includere e per contrastare la povertà. Ora ci sono a disposizione il doppio delle risorse che aveva il vecchio reddito di inclusione, la misura prima prevista per contrastare la povertà. Il reddito di cittadinanza non ha funzionato, perché ha voluto essere una misura per coniugare contrasto alla povertà e politiche attive, ma non c'erano gli strumenti per poterlo fare, innanzitutto per la macchinosità delle procedure previste per il passaggio tra ottenere il reddito di cittadinanza ed entrare nel mondo del lavoro, poi per il fatto che la macchina amministrativa era certamente impreparata a gestirlo. Va detto che i circa 30 miliardi impiegati in quasi quattro anni sono andati in larga parte a famiglie del Mezzogiorno, molti nella mia Campania, in un periodo in cui l'economia ha rallentato, fino a retrocedere duramente dopo la pandemia. Questo ha consentito a molte famiglie di avere un reddito o un'integrazione di reddito che ha sostenuto l'economia di quei territori, però indebitando lo Stato. Ora si cambia pagina e la nuova misura, l'assegno di inclusione, segna un approccio completamente nuovo. Rimangono comunque molte risorse stanziate nel 2024; sono appostati 5,5 miliardi di euro, che andranno ai veri poveri. investono risorse finanziarie nelle politiche attive e sulla formazione, per consentire a chi può lavorare di prepararsi a ricoprire un ruolo attivo nel mondo del lavoro. Il lavoro è quello strumento che dona dignità ed è quel ruolo che ci si conquista nella società, a qualsiasi livello, che fa sentire il lavoratore un cittadino a pieno titolo. Il lavoro e il salario che si percepisce ogni mese tornano a costituire l'autentico reddito di cittadinanza. Ecco perché questo decreto segna un cambio di paradigma rispetto a prima: una visione del mondo inclusiva e non meramente assistenzialista, una concezione della società in cui lo Stato aiuta il cittadino a prepararsi, attraverso la formazione continua, ad ogni nuova sfida, guadagnandosi a pieno titolo il proprio ruolo di cittadino. Allo stesso tempo lo Stato sostiene con un apposito assegno chi rimane indietro, chi è veramente povero e non riesce ad acquistare quei beni materiali veramente necessari a una vita dignitosa. Altro capitolo importante di questo decreto-legge è il proseguimento nella riduzione del cuneo fiscale, iniziata con la prima legge di bilancio del Governo Meloni. Anche su questo l'Esecutivo, con la sua maggioranza, tiene fede al programma elettorale, che non era solo una promessa, ma diventa una realtà, quella di ridurre la pressione fiscale. Dopo aver adottato un aliquota fissa molto bassa per indurre i lavoratori autonomi fino a 85.000 euro di reddito a impegnarsi e a produrre di più, dopo aver approvato un'aliquota fissa molto vantaggiosa per chi inizia a lavorare e per i primi cinque anni, nel decreto prosegue la riduzione delle tasse sul lavoro per i lavoratori dipendenti, portando il vantaggio fiscale rispetto a prima fino a 7 punti percentuali sui redditi fino a 25.000 euro e a 6 punti percentuali sui redditi fino a 35.000 euro. Detto in soldoni, un lavoratore può arrivare ad ottenere in busta paga fino a 100 euro netti in più ogni mese. Dal punto di vista del bilancio pubblico vengono aggiunti altri 4 miliardi di euro ai 3 miliardi già appostati nella legge di bilancio di dicembre. A copertura viene utilizzato integralmente il maggior indebitamento deliberato dalla Camera ad aprile, al quale si aggiungono ulteriori economie di bilancio. La vera sfida è riuscire a trovare le opportune coperture finanziarie per rendere strutturali questi tagli al cuneo fiscale attraverso una maggiore crescita dell'economia e il recupero di evasione delle tasse. Un terzo punto che vorrei sottolineare rispetto alle norme approvate in questo decreto-legge è la volontà di azionare un ulteriore leva a favore dei lavoratori delle aziende private attraverso l'ampliamento del *welfare* aziendale. In questo caso viene concesso l'utilizzo di *fringe benefit* per 3.000 a favore dei lavoratori con redditi bassi per coprire il rincaro delle bollette energetiche. Su questo tema crediamo che si debba fare di più, convinti che il *welfare* aziendale sia non solo un'arma efficace per garantire al lavoratore un reddito netto più alto, ma anche per rendere più armonioso e amichevole il rapporto tra un'azienda e i dipendenti che per essa lavorano. Le aziende che crescono di più sono quelle in cui vengono attivati tutti gli strumenti possibili del *welfare* a favore dei lavoratori. Bene anche la strada intrapresa nel decreto-legge per andare incontro alle esigenze delle imprese che chiedono lavoro flessibile e temporaneo che, essendo contrattualizzato, elimina lo spettro del lavoro nero. Bene gli incentivi per l'occupazione giovanile, che soprattutto nel Mezzogiorno si rileverà una misura utile ed efficace. Si tratta per la vasta articolazione dei suoi diversi interventi agisce in modo puntuale in molti settori, trovando la soluzione più efficace. Forza Italia ha seguito il lungo esame in Commissione e posso testimoniare l'ascolto diligente che si è dato alle istanze di tutte le categorie e la lettura attenta delle modifiche proposte dai Gruppi parlamentari.

giorno in cui il Governo si è riunito per condannare definitivamente i nostri giovani e le future generazioni alla perpetua disoccupazione, firmando un decreto-legge che molto più semplicemente il MoVimento 5 Stelle ha già ribattezzato decreto precariato. Ci aspettavamo l'ascolto delle principali categorie sociali soprattutto per rivedere gli strumenti di ingresso nel mondo del lavoro. Eppure, tutte le audizioni parlamentari sono state più un compitino da dover svolgere in tempi rapidi che un reale banco di confronto. Ci aspettavamo un dialogo schietto, ma concreto tra tutte le forze politiche, nel rispetto dei ruoli di maggioranza e di opposizione. Eppure ci troviamo oggi a discutere un provvedimento che porta solo la firma di chi non sente o meglio non vuole sentire le richieste provenienti dal mondo del lavoro. Dato che ormai questo Esecutivo agisce a colpi di decretazioni di urgenza, ci aspettavamo anche un provvedimento capace di dispiegare effetti in tempi rapidi. L'operatività di queste misure necessiterà invece dell'emanazione di ulteriori decreti attuativi. Ecco, ci saremmo aspettati un maggiore impegno sul tema della riduzione drastica del precariato, della salute, della sicurezza e dei controlli; invece questo decreto-legge è un insulto a tutti quei giovani che vengono quotidianamente umiliati con tirocini fittizi, contratti precari e paghe da fame. Da più parti sentiamo dire che questo decreto-legge porterà ad un taglio del cuneo fiscale e quindi ad un aumento dello stipendio netto in busta paga. Evidentemente però si tratta solo di *marketing* politico, nato per nascondere provvedimenti vergognosi. In realtà, a meno che la misura non venga prorogata ulteriormente, nel Paese questo taglio durerà solo centocinquanta giorni. Onorevoli colleghi della maggioranza, da mesi state urlando che l'abrogazione del reddito di cittadinanza alleggerirà le tasche dello Stato, ma vi chiedo: a danno di chi? Sicuramente degli ultimi, dei fragili, di chi non ha voce, perché evidentemente anziché puntare al recupero dell'evasione fiscale, anziché parlare di tasse come pizzo di Stato, questo Governo ha deciso di fare cassa - o addirittura cresta cresta - sui poveri, su chi a stento riesce a mettere un piatto a tavola e non oso immaginare cosa accadrà nel 2024, quando di fatto entrerà in vigore la revisione del reddito di cittadinanza. Eh già, perché vi siete rimangiati la favoletta propagandistica di eliminare il reddito di cittadinanza per fare posto all'assegno di esclusione. Voi l'avete chiamato assegno di inclusione, ma è paradossale che si chiami così una misura *ad excludendum*,una misura categoriale e non più universale come richiesto dall'Europa e come esiste in Europa. Avete scatenato una guerra ideologica contro i poveri e contro i percettori del reddito di cittadinanza che avete definito furbetti, fannulloni, truffatori, divanisti. È una vergogna. La verità è che il reddito di cittadinanza, misura presente negli ordinamenti di quasi tutti i Paesi europei, ha salvato dalla disperazione milioni di italiani, soprattutto nei durissimi mesi pandemici. Senza questo sostegno, difeso persino dal Commissariato al lavoro dell'Unione europea, avremmo avuto un milione di poveri in più e non lo dico io, bensì l'ultimo rapporto dell'Istat, che fa eco a quanto dichiarato recentemente dal Presidente della CEI. Se solo il Governo fosse stato interessato al corretto funzionamento del reddito di cittadinanza, avrebbe dovuto disciplinare misure drastiche contro i governatori delle Regioni che hanno ritardato le assunzioni nei centri per l'impiego *(Applausi)*, motivo per cui abbiamo presentato un emendamento volto ad accelerare le assunzioni nei centri per l'impiego, prevedendo il commissariamento delle Regioni che non hanno speso le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2020. Questa maggioranza ha ignorato totalmente i nostri emendamenti a tutela dei più fragili e di chi rischia di rimanere indietro, come la mia proposta di prorogare fino alla fine dell'anno lo *smart working* per i lavoratori fragili, giacché tale diritto scadrà il prossimo il prossimo 30 giugno. Avete approvato un emendamento per prorogare il lavoro agile, ma solo per i privati e nel pubblico zero. La motivazione è che non siamo in grado di stabilire la platea dei potenziali fruitori. Ma come? Non eravate pronti a governare? E ora non sapete quanti sono i fragili, gli immunodepressi, i malati di cancro o i trapiantati? Vergognosa, ad esempio, è la previsione di rafforzare la possibilità di ricorrere anche ai contratti a termine, un chiaro regalo a quei datori di lavoro che eludono che eludono il sistema sfruttando milioni di lavoratori e che in tal modo potranno prolungare questa forma contrattuale alimentando la precarietà in Italia. La previsione secondo cui i datori possono assumere fino a due anni senza causali ad eccezione di motivazioni di natura tecnica, organizzativa e produttiva, disciplinate o da disciplinare, aumenterà secondo noi il contenzioso giudiziario e questo perché in assenza di una disciplina contrattuale la causale verrà definita in autonomia dalle parti del contratto, incrementando la condizione di già forte debolezza di tanti lavoratori. Inoltre, avete aumentato il tetto per i *voucher* e in questo modo i *voucher* prenderanno il posto dei regolari contratti di lavoro, un insulto a migliaia di lavoratori soprattutto stagionali. Voglio ricordare che già con la legge di bilancio 2023 il Governo Meloni era intervenuto per modificare le prestazioni di lavoro occasionali, prevedendo l'aumento da 5.000 a 10.000 del 10.000 del limite massimo dei compensi da corrispondere, un chiaro segnale di sostegno al mondo della precarietà, confermato dai recenti dati dell'osservatorio sul precariato INPS, secondo cui il numero dei lavoratori impiegati con contratti di prestazione occasionale è in aumento. Cari concittadini - è a loro che mi rivolgo oggi attraverso il suo tramite, signor Presidente, perché i senatori e le senatrici sono stati sordi ai nostri emendamenti - abbiamo provato a modificare questo decreto presentando numerose proposte di buonsenso nell'interesse unico dei nostri veri datori di lavoro: i 60 milioni di italiani. Eppure spiace evidenziare che tutte le proposte del MoVimento 5 Stelle sono state stralciate probabilmente perché dirette ai lavoratori e non agli sfruttatori a cui il Governo strizza invece un occhio. *(Applausi)*. Penso alla bocciatura di un nostro emendamento volto a introdurre nel nostro ordinamento il salario minimo non inferiore ai 9 euro lordi un'iniziativa appoggiata dalla stessa Commissione europea. Penso a una mia proposta emendativa che intendeva introdurre un'indennità in caso di violenza di genere per le lavoratrici autonome. Penso alla decontribuzione totale per i contratti di lavoro domestico, una proposta voluta fortemente per valorizzare un settore tanto delicato quanto vitale a livello economico e sociale. inoltre al fondo per la competenza digitale, volto a contrastare il divario digitale e culturale e per sostenere la massima inclusione, favorendo l'educazione sulle tecnologie del futuro. Insomma tagliola, a cui già ci ha abituato il Governo Meloni, questa volta si è abbattuta sulle nostre richieste di modifica, incrementando ancora di più il divario tra ricchi e poveri, tra occupati e disoccupati. Pertanto, innanzi a questo provvedimento che ignora totalmente i profondi cambiamenti del mercato del lavoro, forti dell'appoggio e della comprensione dei 20.000 manifestanti a Roma che il 17 giugno hanno gridato "no alla precarietà", qui ribadiamo con forza il no alla deriva pericolosa del Governo Meloni e di una destra a-sociale - che vuole sempre più convincere il popolo italiano che la povertà sia una colpa. Ma noi non lo consentiremo.

di cui mi occupo, il provvedimento in discussione, al Capo II, contiene alcune lodevoli disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro orientate allo sviluppo delle misure di prevenzione e di protezione, in particolare di carattere organizzativo-gestionale, dove sicurezza è sinonimo di salute, e per il rafforzamento delle regole - già esistenti - di tutela contro gli infortuni, così come per il potenziamento dei controlli ispettivi in tutto il Paese, con previsioni atte a supportarne l'osservanza applicativa per un migliore governo dei rischi secondo le specificità aziendali. Così agendo in effettiva formazione e competenza datoriale in materia di sorveglianza sanitaria e attività del medico competente, nonché con l'integrazione e la condivisione dei dati e delle informazioni disponibili per una programmazione sempre più incisiva e mirata dei controlli ispettivi, soprattutto in chiave preventiva e deflattiva. Dobbiamo infondere la cultura della sicurezza e questo provvedimento va nella giusta direzione. Si tratta di marginalizzare quelle aree grigie dove si formano fattispecie generatrici di incidenti essenzialmente per inerzie e distorsioni legate ad inadeguatezze, concausa di gran parte degli infortuni, per non essere più "distratti" in ordine all'applicazione di procedure di sicurezza note e consolidate da tempo, quando il vero tema è proprio, puramente e semplicemente, il loro rigoroso rispetto. Certo ciò non è scontato, soprattutto perché spesso taluni accorgimenti vengono disattesi proprio dagli stessi addetti per eccesso di confidenza con gli strumenti utilizzati. Apprezzabile attenzione viene inoltre posta alla tutela degli studenti in formazione, non solo quanto alla loro copertura assicurativa INAIL, ma anche creando un fondo che che preveda il ristoro delle famiglie degli studenti in formazione vittime di infortuni (anche se questo non dovrebbe più succedere). Credo sia un segnale positivo perché il principio è lo stesso, anche per finalmente riconoscere il giusto ristoro ai medici vittime del Covid e - se deceduti rimasti in assenza di qualsivoglia tutela in forma assicurativa. La sfida è coniugare sicurezza, salute, lavoro ed impresa, agendo per andare oltre il mero controllo ispettivo e il mero approccio ispettivo e prettamente sanzionatorio, posto che senza competitività non c'è futuro, non c'è mercato; senza mercato, non c'è impresa; senza impresa, non c'è lavoro. Senza lavoro sicuro e latore di salute non ci sono né crescita, né sviluppo, perché quando c'è un infortunio sul lavoro di una certa gravità, fino ad arrivare a quelli mortali, i costi umani e sociali sono inaccettabili; tuttavia, è altrettanto vero che i costi economici, anche a carico dell'impresa, sono molto pesanti. Siamo consapevoli che in taluni settori (l'edilizia è uno fra questi, come noto l'anno scorso è stato il settore che ha avuto più infortuni mortali) tutto è più complesso, perché in molti si improvvisano. Pertanto la formazione e l'addestramento specifico, così come previsto dal decreto-legge, a carico del datore di lavoro che utilizza personalmente apparecchiature che richiedono conoscenze particolari, intende incidere proattivamente sul cambiamento di rotta, a garanzia di adeguata, essenziale conoscenza e competenza datoriale. L'orizzonte a cui tendere è un sistema evoluto ed integrato di prevenzione, sicurezza e salute, tanto nell'impiego che nella realizzazione dei prodotti, a cominciare da quelli di nuova immissione sul mercato. Al riguardo entriamo in un mio *mantra,* quello della prevenzione predittiva, perché, come molti di voi sapranno, all'inizio dell'introduzione su base volontaria della certificazione di qualità, molti storcevano il naso perché la consideravano un costo. Ebbene, i dati sono lì a dimostrare che la qualità è un ricavo, così come lo sarà investire strutturalmente in governo dei rischi e in sicurezza. Ovviamente, di questi tempi tutti ci occupiamo di risparmi energetici perché lo *shock* che stiamo ancora superando (e non è detto che lo sia) è tale che per molto tempo si parlerà di rinnovabili, di immobili meno energivori e di tutto il corollario. Pertanto, il pensiero prevalente è quello di risolvere quel problema, che deve essere ricondotto nella transizione energetica mediante, per esempio, l'impiego di materiali da costruzione tali per cui le case del futuro siano decisamente meno energivore, antisismiche e non rilascianti inquinanti a vario titolo. Cosa voglio dire? Negli anni Sessanta l'amianto era usato diffusamente, senza aver fatto le dovute preventive verifiche sulla garanzia di salubrità del materiale. Dobbiamo quindi imparare dal passato ed errori simili non si devono più ripetere; pertanto, anche per materiali che sembrano molto promettenti si devono fare delle istruttorie molto approfondite, affinché ciò che oggi, anche solo per moda o per tendenza, appare interessante non si dimostri in futuro ad elevata incidenza di rischio per la salute e per l'ambiente. Dobbiamo imparare a vedere nelle nuove tecnologie l'opportunità per cambiare paradigma; tuttavia, proprio perché dobbiamo farlo e proprio perché si tratta di nuove tecnologie e di nuovi prodotti, dobbiamo far sì che già dalla progettazione vi sia una maggiore sicurezza intuitiva sul lavoro, sia per le imprese che li realizzano, sia per le aziende che andranno ad impiegarli, e una maggiore sicurezza a tutela della salute individuale e collettiva, non solo nella produzione, ma soprattutto nell'utilizzo. Vorrei essere ancora più esplicita: non dovremmo permettere, non solo per gli alimenti e i mangimi sintetici, che possa entrare sul mercato un nuovo prodotto, se non vi è una chiara e e documentata evidenza scientifica di prevenzione di ogni possibile rischio, financo con prove palesi di accelerato invecchiamento, posto posto che il produttore dovrebbe dimostrare non solo di avere a cuore la sicurezza degli operatori che lo realizzano, ma soprattutto la salute di chi lo andrà ad utilizzare. Siamo consapevoli che il contributo di questo provvedimento è solo un primo passo, ma in linea con un cambio di prospettiva dove tanti, anche piccoli, piccoli, primi passi - e anche se ogni tanto c'è un passo di lato, ma vi porremmo sicuramente rimedio - contribuiranno a far sì che vi sia un sistema lavoro sempre più proattivamente sicuro e salubre.

che aveva assicurato al suo primo incontro presso la Commissione competente per questo decreto-legge la sua presenza, la sua partecipazione e una grande volontà di confronto. Si sa che le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni. Poche cose quanto il valore del lavoro, il suo ruolo per l'individuo e per la società da un lato e, dall'altro, poche cose quanto la povertà (laddove non sia una scelta personale, magari per ragioni religiose, ma una condizione esistenziale) possono segnare tanto la distanza tra differenti culture politiche. Lo abbiamo toccato con mano, se avevamo bisogno di un'altra prova, proprio con questo decreto-legge, che non contrasta la povertà, ma combatte i poveri. Un decreto-legge che ha come titolo vero "precarietà e povertà" e che noi continueremo a chiamare così. I dati presentati ieri dall'Ufficio parlamentare di bilancio hanno fotografato gli effetti che devasteranno la vita di questi poveri e che derivano dalla sostituzione del reddito di cittadinanza con questo assegno di inclusione. Probabilmente - immagino - è da qui che è derivata la volontà di presentare in Aula, da parte della relatrice, un emendamento che cambia la misura di equivalenza, perché avete dovuto prendere atto che questi dati, presentati da un organismo assolutamente terzo, ci dicono che cento è la percentuale che riguarda le famiglie e -28 per cento sono le risorse che andranno a contrastare la povertà, il che dimostra che combatte i poveri e non la povertà. Il decreto è innervato da un pregiudizio e questo mi ha molto colpito, devo dirvi, al di là delle appartenenze politiche. Sono rimasta colpita dalla pochezza - non me ne vogliano i colleghi - del confronto in Commissione, dove questo testo è approdato oltre un mese fa, una pochezza che rattrista: sentire parlare solo di gente che non ha voglia di lavorare e che sta sul divano è davvero Questo decreto - come vi dicevo - è innervato da un pregiudizio ed è per questo che ho parlato di cultura politica: questo pregiudizio afferma che la povertà è uno stato di colpevolezza.

che comprendo in parte; ci si sottrae sempre, quando si è in maggioranza, a un confronto vero, perché è più facile, si scappa dalle cose, però non va a finire bene di solito e poi si cambia idea e ci si deve correggere.

che in questo decreto perde il valore straordinario che gli è assegnato dalla Costituzione, all'articolo 1 e all'articolo 4, ed è così che perde dignità. Hanno scritto due studiosi per la rivista "Il Mulino" che «Quello che si prospetta di fronte a noi non è, dunque, solo un imperdonabile, cattivo,

sempre meno tutelati», come hanno detto le mie colleghe benissimo, e non torno su questo punto. Siamo davvero di fronte all'impossibilità di «garantire una vita dignitosa e decorosa. Contrastare questa misura è, tra le altre cose», come scrivono ancora questi due studiosi, «nell'interesse di chi difende il valore della dignità del lavoro». Facendo così, queste norme non corrispondono in alcun modo al dettato costituzionale, laddove all'articolo 36 i padri costituenti hanno affermato che «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»: libera dal ricatto e dignitosa, come è diritto di ogni essere umano. Il decreto divide i poveri tra i meritevoli, che hanno non autosufficienti o minori a carico, e i non meritevoli, che non hanno invece questi carichi. Così facendo, lo si trasforma in una misura categoriale, ed è questo uno dei *vulnus* più gravi del decreto in esame, perché questo è un errore che, in parte, abbiamo tentato inutilmente di correggere: è la negazione della necessità dell'universalità. Una misura che davvero di contrasto alla povertà deve essere per sua stessa natura universale e, di fatto, in tutti i Paesi europei esiste una misura di sostegno al reddito rivolta ai poveri. Il Consiglio europeo, proprio di recente, ha varato una raccomandazione a favore di un sostegno al reddito, mediante appunto un reddito minimo. Quindi, continuiamo ad andare in una direzione che ci porta lontano dai Paesi europei

ha ricordato Annamaria Furlan, si deve andare a qualunque distanza, magari con un *part-time* e, se non si rispettano le regole, se un componente della famiglia che viene considerato occupabile non segue tutte queste regole, il nucleo familiare nel suo insieme perde il reddito, negando tra l'altro anche i diritti dei minori. Gli esperti hanno inutilmente segnalato sono ben pochi i centri per l'impiego in grado davvero di accompagnare i beneficiari nei termini previsti dal decreto, termini in questo caso cronologici, di tempo. Le norme

ciò che è necessario quando si vuole accompagnare e fare uscire dalla povertà chi è in stato di bisogno. Sappiamo che il reddito di cittadinanza aveva dei difetti, non ho nessun problema a dirlo, che andavano corretti. D'altra parte, proprio per iniziativa del Partito Democratico, venne introdotta per la prima volta una misura universale di contrasto alla povertà. Si trattava del reddito di inclusione

*magna pars* la presenza della Lega, che oggi sembra avere completamente dimenticato di essere tra coloro che hanno votato il reddito di cittadinanza e partecipato ai festeggiamenti per la sua approvazione. *(Applausi)*. Noi non smetteremo però di ricordarvelo, quindi preparatevi, perché ogni volta che prenderò la parola andrò a vedere che cosa ha fatto la Lega nel Governo Conte I, che cosa ha fatto nel Governo Conte II e anche nel Governo La logica del decreto, come dicevo, sembra derivare dalla congiunzione tra un giudizio negativo sulle politiche contro la povertà e una priorità attribuita alla natalità e anche in questo è destinata evidentemente a fallire. In sostanza, il messaggio che arriva è che, se si è poveri, lo Stato non è disposto ad assicurare un sostegno per vivere decentemente. Non posso

come è ovvio, e con esso concordati. Si tratta di emendamenti rispetto ai quali la Commissione bilancio non ha ancora potuto esprimersi in assenza delle relazioni tecniche. tentativo per rimediare al gravissimo errore compiuto dalla ministra Calderone, che ha tagliato del 50 per cento il fondo per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

alcune sono state dette con grande positività, altre con un fare che io ho trovato costruttivo. Si è parlato di indifferenza del Governo Meloni, di arroganza, di esaltazione esaltazione della precarietà, di un tentativo e di una voglia di colpire i poveri, di aumentare le disuguaglianze; si è parlato di provvedimento vergognoso, addirittura di cresta sui poveri, di lotta ideologica; di dividere il sistema tra lavoratori e sfruttatori. Si è detta una serie di parole, che però non fanno il paio con una realtà con la quale dobbiamo confrontarci, una realtà che pone in evidenza una parola che non è stata mai pronunciata in questo dibattito: la parola è "sostenibilità". Tutto il sistema dell'inclusione sociale e lavorativa può andare avanti e può produrre frutti, se il sistema Paese si sostiene,

piazze, ma nel sacrificio e nel lavoro che il nostro *premier* Giorgia Meloni sta compiendo nel mondo intero, tenendo alta la credibilità e l'affidabilità della nostra Nazione, dell'Italia,

quanto il nostro Stato è capace di attrarre investimenti. I dati che ci dicono che siamo sulla strada giusta sono lo *spread*, che è a livelli minimali (considerate quanto questo rende al nostro Stato), e il PIL, che si La sostenibilità, come detto, è un discorso che fa il paio anche con un PIL che si innalza. E questo PIL si innalza perché vengono esaltati alcuni settori produttivi che trovano il proprio sostentamento nelle misure che noi e il Governo abbiamo introdotto in questo decreto-legge, decreto-legge, quelle che voi chiamate misure di precarietà, quando invece sono misure importanti per coniugare domanda e offerta di lavoro in alcuni settori particolari che non possono e non riescono a determinare una stabilità del lavoro per la loro specificità e non per la loro volontà. Dovremmo sostenere le misure che, per esempio, il ministro Santanchè e il ministro Sangiuliano stanno portando avanti per destagionalizzare il turismo o che il ministro Lollobrigida sta portando avanti una protezione e una valorizzazione del *made in Italy* e dei nostri prodotti agroalimentari, che possono determinare la stabilità del lavoro. La seconda parola che è mancata e che invece noi citiamo molto spesso è resilienza. Che significa resilienza? È la capacità di affrontare momenti di crisi venendone fuori più forti. È questo che vogliamo noi in tutte quelle persone che vogliamo includere nell'inclusione sociale e lavorativa: fare in modo che in loro si accresca la capacità di affrontare la crisi e la la condizione in cui versano, per poterne uscire più forti. Questo concetto di rafforzamento coinvolge sì la collettività, ma coinvolge soprattutto i singoli. Perché ne devono uscire più forti? Ne devono uscire più forti perché la la si ritrova nel lavoro. La dignità non si ritrova in un messaggio subliminale che arriva alle persone,

Quando la collega Zampa parlava di un collega che in Commissione ha citato la parola sacrificio, quel collega ero io. io. La ringrazio, collega Zampa, perché la parola sacrificio in questo dibattito l'ha citata solo lei, prima di me. La cito e la valorizzo io, ora, perché, quando una sua collega - mi pare Furlan - parla di ascensore sociale, l'ascensore sociale su che cosa si è fondato se non sul sacrificio? In Commissione In Commissione si è detto che addirittura noi produciamo nuovi schiavi, perché schiavizziamo quelle persone che perdono il beneficio se solo non accettano un lavoro a tempo indeterminato sul territorio nazionale o a tempo determinato entro i limiti di 80 chilometri o di 120 minuti di percorrenza con i mezzi pubblici. Se queste persone non accettano e perdono il beneficio, le abbiamo schiavizzate. E allora io vi chiedo: chi è più schiavo, quella collettività che attraverso il sacrificio e attraverso la tassazione trova la copertura di spesa per determinare misure di inclusione sociale oppure qualcuno che, sulla base di sacrificio, non riesce ad accettare queste condizioni? Così facendo, a mio avviso, lo schiaffo lo dà non a noi di maggioranza, ma a tanti nostri padri e a tanti nostri nonni, che con sacrificio hanno dovuto emigrare oltre i confini nazionali per dare dignità a se stessi, alle loro famiglie e al lavoro. C'è un dato ineludibile che noi dobbiamo tenere presente.

Tale comma afferma che «Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società». Voglio citare Aldo Moro, il quale diceva che questo Paese non si salverà, che la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera, se in Italia non nascerà un nuovo senso del dovere. Noi vogliamo che la stagione dei diritti e delle libertà non sia effimera perché dobbiamo capire che abbiamo tutti il dovere di concorrere alla crescita e alla sostenibilità del nostro Paese. Vogliamo coniugare libertà, doveri e diritti e lo facciamo guardando all'inclusione sociale e lavorativa e valutando le potenzialità di accesso al lavoro. Non si è detto che si discrimina o si creano diseguaglianze tra chi ha accesso al lavoro; non è vero, non corrisponde a verità. L'accesso al lavoro è condizionato da un piano individualizzato di valutazione per le potenzialità che una persona può e

Voi avete una visione parziale del mondo del lavoro, noi pretendiamo e pensiamo di avere una visione globale del mondo del lavoro, che parte da una necessità essenziale: la sostenibilità del nostro Paese e del sistema delle nostre imprese, ma anche la valorizzazione delle relazioni sindacali e delle norme di igiene e sicurezza del lavoro che possono permettere il benessere psicofisico, ma anche economico e di miglioramento della qualità di vita del lavoratore e delle loro famiglie, e la ricaduta in termini di crescita civile e sociale del nostro Paese. Ecco, questa è la visione che noi abbiamo voluto

certamente chi ha mostrato oggi in quest'Aula degli atteggiamenti propositivi nei confronti di tale riforma a cimentarsi con noi per trovare delle soluzioni strutturali, soluzioni strutturali, vantate e chieste per il cuneo fiscale che noi abbiamo introdotto e portato fino al 31 dicembre - mai avvenuto finora - che anch'esse ad una crescita della nostra collettività e della sostenibilità.

lavoratore e il miglioramento delle norme di igiene e sicurezza del lavoro, intendono creare e avviare un percorso di miglioramento della qualità di vita dei lavoratori e delle loro famiglie.

intendo esprimerle e significarle tutto il disappunto del mio Gruppo, il MoVimento 5 Stelle, per questo slittamento dei lavori che dimostra davvero la mancanza di rispetto per i lavori di questa Assemblea. Questo ritardo è dovuto a

emendamenti della stessa relatrice vengono presentati all'ultimo secondo, mancanti della necessaria relazione tecnica del MEF, provocando il ritardo dei lavori di questa Assemblea e mancando quindi di rispetto alla stessa. Mi permetto di aggiungere un'altra notazione: ancora una volta si è replicato il costume che questa maggioranza ha sviluppato e messo in piedi di bocciare emendamenti proposti dalle opposizioni per poi farli propri e riproporli come emendamenti propri o addirittura in forma di decreto-legge. *(Applausi)*. Poiché noi abbiamo sempre predicato la condivisione, abbiamo sempre detto che siamo disponibilissimi a collaborare, se ci volete copiare, copiateci, ma almeno chiedete il permesso, non fatelo con questi metodi autoritari tipici di questa maggioranza.

fare una precisazione al senatore Magni. Innanzitutto, l'articolo che riguarda la scala di equivalenza è assolutamente comprensivo di una relazione illustrativa e tecnica precisa e puntuale e quindi questo mi sembrava doveroso precisarlo. Inoltre, mi risulta assurda la sua polemica circa la presentazione di un mio emendamento, se la necessità è proprio quella di porre ulteriori somme per quello che riguarda la sicurezza sul lavoro e soprattutto gli infortuni mortali, quindi veramente sono polemiche sterili che da relatore di un decreto-legge che ritengo così importante lasciano il tempo che trovano.

e quindi se fosse possibile, anche per un'interlocuzione che abbiamo avuto con i colleghi senatori delle opposizioni che chiedevano degli approfondimenti con alcune note che sono appena arrivate dal MEF, saremmo pronti intorno alle ore 14. Se lei decide di sospendere la seduta, a noi serve una mezz'ora di tempo per poter valutare tutta la parte degli emendamenti della relatrice e alcuni subemendamenti che sono arrivati. Dopodiché, per le ore 14 potremmo essere pronti per iniziare a votare.

mese. Abbiamo dovuto assistere al deposito di emendamenti della relatrice ieri e oggi, con la necessità quindi di uno slittamento dei lavori per consentire alla Commissione bilancio di intervenire oggi, nonostante avessimo deciso tutti insieme che la seduta sarebbe continuata dalle ore 13 per il voto sugli emendamenti. Secondo noi questo è un modo di procedere non molto rispettoso delle opposizioni, anche perché ricordo che tali emendamenti sono stati depositati ed è stato dato un termine ridicolo per la presentazione di subemendamenti, quindi è stato dato anche molto poco tempo per esaminarli. Tenuto conto del fatto che si tratta di un provvedimento importante e sul quale la Commissione ha lavorato a lungo, riteniamo inaccettabile questo modo di procedere e siamo totalmente contrari alla sospensione dei lavori.

La seduta è ripresa.

l'immediata convocazione della Conferenza dei capigruppo, intanto perché ci sono temi regolamentari che abbiamo il dovere di affrontare in quella sede. Abbiamo Abbiamo trovato non solo fuori luogo, ma anche abbastanza goffa la spiegazione del Presidente della Commissione bilancio e non solo perché eravate arrivati al novantanovesimo cancello e siete tornati indietro, ma perché, come lei sa, signor Presidente, per la sua esperienza parlamentare, non esiste il voto pari: quando si è pari, vuol dire che l'emendamento è stato respinto. Quindi, o si è pari, o si è inferiori alla parità, quando c'è una votazione, se non c'è un voto in più, chiunque viva le Aule parlamentari

e alla fine il risultato è stato quello che è sotto gli occhi di tutti: sono stati bocciati tutti gli emendamenti presentati oggi dalla maggioranza. Come lei sa, signor Presidente non è possibile riproporli

rammendi peggiori dei buchi, pretendendo poi di andare avanti come se nulla fosse successo. Non ve lo permetteremo. Pretendiamo il rispetto delle regole. Per questo, signor Presidente, chiediamo la convocazione della Conferenza dei Capigruppo e chiediamo che le Commissioni di merito, innanzitutto la 10a Commissione e la Commissione e la Commissione bilancio si riuniscano successivamente alla Conferenza dei Capigruppo per tornare ad analizzare il testo, che non potrà più comprendere gli emendamenti che oggi sono stati bocciati. Signor Presidente, colleghi, posto che non mi affascina tanto il gioco per cui, quando si è maggioranza, si ragiona in un modo e, quando si è opposizione, si ragiona in un altro, dico che oggi c'è però un elemento nuovo, molto innovativo, che non ha precedenti. Mi riferisco al fatto che in Commissione bilancio la maggioranza è andata sotto sull'approvazione del parere che la Commissione dà all'Assemblea sugli emendamenti. Questa è una cosa che non ha precedenti: quindi, dopo il DEF che non aveva precedenti, un'ulteriore innovazione di precedenti da parte di questa compatta maggioranza *(Applausi)* sul tema dei pareri della Commissione bilancio. Credo che per questa ragione e, soprattutto, per la gestione dei tempi, da adesso in poi sia necessaria la Conferenza dei Capigruppo. Il presidente Calandrini ha semplicemente detto un'ovvietà: si cambia il parere. Posto che per il noto principio del *ne bis in idem* non si può votare di nuovo lo stesso parere, ci sarà un parere che su un emendamento verrà modificato e si rivoterà il parere. Credo, tuttavia, che il dato politico e anche il rapporto tra maggioranza e opposizione ci consentano di chiedere come forza di opposizione la convocazione della Conferenza dei Capigruppo per gestire i tempi con i quali arriveremo al voto finale su questo decreto-legge. Lo dico con un po' di amarezza perché, nonostante il tentativo encomiabile del presidente Zaffini in Commissione, ricordo che gli emendamenti segnalati sono stati depositati il 28 maggio, il 28 maggio, quasi un mese fa. La maggioranza e il Governo non sono riusciti a costruire il loro percorso emendativo su un testo che stava lì da un mese

Evidentemente non si è in grado di fare un lavoro ordinato e quindi ritengo che sia la Conferenza dei Capigruppo a dover affrontare la questione.

Presidente, vorrei rammentare il fatto che questo decreto-legge è stato annunciato con una propaganda di stampa che diceva che sarebbe stato il più grande taglio del cuneo di tutti gli ultimi anni. Non siete stati in grado nemmeno di garantire la maggioranza per il più grande taglio del cuneo degli ultimi anni. E questo è un problema. Vedete, chi vi parla non ha un atteggiamento ideologico su questo decreto; ne vede i lati buoni e i lati meno buoni. Il punto è politico: politico: non siete in grado, all'interno delle Commissioni, di garantire la maggioranza neppure per le cose per le quali fate una propaganda esasperata nel Paese. Ve lo dico in modo molto chiaro: nonostante una posizione che è molto articolata sui temi del decreto, noi ci associamo alla richiesta di convocazione della Conferenza dei Capigruppo fatta dagli altri colleghi dell'opposizione *(Applausi)*, perché è del tutto evidente che la riprogrammazione dei lavori dell'Assemblea deve essere fatta sulla base di quello che è avvenuto e che non si possa fare finta di nulla. potete anche aver fatto un'operazione parziale sul taglio del cuneo, ma di sicuro non siete in grado, nei lavori delle Commissioni, di portare avanti nemmeno il minimo lavoro che impostate. È successo un fatto grave, che non può essere declinato come una non maggioranza, come ha detto il presidente Calandrini, che rispetto e che è persona seria. Peraltro ricordo Peraltro ricordo a tutti che la parità è stata raggiunta con il voto del presidente Calandrini; questo in qualche modo dovrebbe spiegare le difficoltà che avete. Non è nostro dovere garantirvi la maggioranza; c'è bisogno di una riprogrammazione dei lavori in Conferenza dei Capigruppo. Quindi, Presidente, la prego di convocarla immediatamente, perché abbiamo tutti bisogno di fare chiarezza. *(Applausi)*.

la settimana scorsa abbiamo fatto una serie di sedute, con riconvocazioni praticamente *ad horas* o anche a minuti, e ogni volta mancavano i pareri o c'erano problemi sugli emendamenti della stessa maggioranza. Quello che è successo in Commissione è davvero grave, ma soprattutto significativo, e certamente non è rispettoso del ruolo di questo Senato pretendere una riconvocazione a mezz'ora, quando si sa che mezz'ora non basterà. La maggioranza deve saper gestire i suoi tempi d'Aula e le sue votazioni e garantire che i suoi provvedimenti arrivino firmati, con i pareri e con i voti necessari per essere portati in Aula. Quindi mi associo alla richiesta di convocazione della Conferenza dei Capigruppo, perché è necessario, nel rispetto di tutti noi, che i lavori vengano calendarizzati tenendo conto di tutto quello che è successo. Presidente, vorrei precisare una cosa che mi sembra superflua, ma che evidentemente non lo è. Siamo tutti ben

era un parere su una serie di emendamenti e ciò non significa assolutamente che questi emendamenti siano stati bocciati. È stato bocciato (nel senso di non approvato) il parere sugli emendamenti. *(Applausi)*. ci sono state due richieste di convocare la Conferenza dei Capigruppo e una richiesta di non farlo, da parte dell'opposizione. Ebbene, io mi rimetto alla decisione del Presidente, ma, per conto del Gruppo Fratelli d'Italia, del tutto superflua una Conferenza dei Capigruppo per una questione che

Senza però perdere tempo, forse è meglio che la Commissione bilancio si ritrovi subito e non alle 15 o alle 15 meno un quarto, e faccia queste valutazioni. Quindi o ci sono effettivamente le condizioni e si è in grado di esprimere un parere sulla base di termini regolamentari chiari e certi

stanno aspettando il provvedimento perché devono avere la tempistica necessaria, al netto di tutte quelle che possono essere le valutazioni politiche. La Conferenza dei capigruppo cosa può chiarire se non semplicemente fare un po' di di grancassa di una situazione che è accaduta? Da un punto di vista regolamentare penso possa essere poco produttiva. le valutazioni affrontando gli emendamenti, la discussione e le dichiarazioni di voto. È semplicemente per cercare insieme una gestione ordinata dall'Aula ribadisco - al netto delle valutazioni politiche che sono evidenti. Sono in maggioranza, lo riconosco e non ci nascondiamo certamente dietro a nessuno. Presidente, mi rivolgo ai miei colleghi per il suo tramite, come si fa in questi casi, non è che qui si sta facendo una pantomima, un gioco delle parti tra maggioranza e opposizione, altrimenti diventa veramente una ridicolizzazione dell'Assemblea, della Commissione e anche delle questioni politiche francamente, almeno dal mio punto di vista, assolutamente non condivisibili. Qui c'è semplicemente un

è anche un po' l'epilogo di una scelta che si è fatta in tutte queste settimane. Tra l'altro, l'Aula era inevitabilmente un po' deserta stamattina,

su come è stato condotto l'*iter* del provvedimento e anche sull'atteggiamento che il Governo ha avuto nei confronti di diversi emendamenti dell'opposizione che, come spesso accade, sono stati messi da parte e poi bocciati senza una motivazione di alcun genere. È evidentemente anche questo il frutto inevitabile della scelta che è stata fatta in tutte queste settimane. Come è stato ricordato, gli emendamenti sono stati presentati molte settimane fa e ricordiamo anche che questo decreto

dal mio punto di vista anche della strumentalità, perché contiene misure che non vanno nella direzione della festa dei lavoratori e delle lavoratrici. In ogni caso, stando ai fatti, si è prodotto un fatto politico all'interno della Commissione. Dopo varie settimane in cui il Governo ha avuto un determinato atteggiamento nei confronti degli emendamenti, anche quelli di buonsenso, presentati dall'opposizione, si produce in Commissione un fatto politico che - la potete raccontare come volete - è un fatto politico evidente: un emendamento che viene proposto in Commissione e che non passa, è bocciato. Non ci sono giri di parole da fare su questo: l'emendamento è respinto. Da questo punto di vista, il Regolamento è chiarissimo, come è chiarissimo quello che è successo negli ultimi cento anni di storia del Senato e quindi mi pare evidente che rispetto a un fatto del genere come minimo bisogna consentire alle forze dell'opposizione che lo stanno richiedendo

però, che è proprio l'epilogo inevitabile di una scelta che è stata fatta in tutte queste settimane. È chiaro che se si sceglie la strada della propaganda e di non confrontarsi nel merito, questo è il frutto inevitabile di un meccanismo tutto sbagliato. sono intervenuto per primo in Aula questa mattina alle ore 10,25 circa in

vi siete dimenticati da un pezzo. *(Applausi. Commenti)*. Ci pensiamo noi oggi ai lavoratori e al lavoro, con l'approvazione di questo provvedimento. che è accaduto in Commissione dal punto di vista politico non ha alcuna rilevanza. Se oggi siete attaccati a questi piccoli episodi non avete argomenti politici per controbattere alla maggioranza.

di soli quindici minuti, quindi io e il senatore Lotito, componenti della Commissione bilancio, sempre presenti al 100 per cento in Commissione, siamo arrivati un quarto d'ora in ritardo. Non c'è alcun problema politico, non c'è bisogno di alcuna Conferenza dei Capigruppo. Possiamo ritornare in Commissione bilancio - perché l'emendamento non è stato votato in maniera contraria

dell'opposizione le respingo. Noi siamo pronti. Invito il Presidente di questa Assemblea a riconvocare anche una Commissione bilancio per tornare a votare. Non c'è nessuna polemica su quello che è accaduto; si è trattato coincidenza di tempi che non c'è stata rispetto a un impegno di Gruppo che avevamo.

per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 13.0.100, 16.0.1, 18.0.1, 19.0.3, 19.0.4, 22.0.1, 23.0.1, 24.0.14, 27.0.1, 27.0.2, 36.101, 38.0.6, 38.0.8, 38.0.14, La Presidenza dichiara altresì inammissibile il subemendamento 25.0.1000/1.

impegna il Governo: a valutare la possibilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica e con l'ordinamento comunitario, di prevedere nel primo provvedimento utile l'applicazione di un'aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni rese alle Agenzie per il Lavoro da enti e società di formazione, finanziati attraverso il fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,

defiscalizzazioni, le aziende private che, per i sei mesi successivi al rientro sul posto di lavoro, avviino percorsi di formazione e crescita delle competenze per le lavoratrici madri nei limiti delle risorse disponibili.

l'assurdità del parere contrario su questo emendamento, che chiedeva solo di estendere alle famiglie con figli al di sotto dei ventisei anni, che quindi stanno facendo un percorso di studi, la possibilità di accedere all'assegno di inclusione. Forse, infatti, la maggioranza e il Governo non si sono resi conto che gli studenti in Italia concludono il ciclo di istruzione secondaria superiore di secondo grado all'età di diciannove anni; voi gli state togliendo il sostegno un anno prima della conclusione degli studi, dicendo che devono andare a lavorare per dare una mano a mantenere la famiglia, a fare gli schiavi, invece che formarsi in un percorso di studi e magari proseguire anche all'università. Ai nostri giovani state dicendo che devono restare ignoranti per fare gli schiavi nelle imprese dei vostri amici. Ditelo ai cittadini italiani quello che pensate veramente.

i commi 4 e 4-*bis* sono sostituiti dal seguente: «4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza: a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni; c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5; d) di 0,3 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione; e) di 0,1 5 per ciascun minore di età, fino a due; f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo. *Conseguentemente*: All'articolo 13

Signor Presidente, ho chiesto la parola per dichiarazione di voto perché il nostro Gruppo voterà a favore di questo emendamento, l'unico tra gli emendamenti e subemendamenti che sono stati presentati Noi prendiamo atto che la maggioranza ha avuto un importante ravvedimento. Dopo Dopo discussioni davvero inutili e superflue in Commissione, credo sia stato molto convincente quanto ieri l'Ufficio parlamentare di bilancio ha diffuso, facendo una fotografia di ciò che avverrà con la sostituzione del reddito di cittadinanza con l'assegno di inclusione: meno 42 per cento sarebbero state, nella prima versione, le famiglie

vorrei fare riflettere la maggioranza sul fatto che questo emendamento avrebbe lo scopo di ancorare l'offerta formativa, i tirocini e quant'altro al territorio in cui vengono erogati. Faccio un esempio: fare un corso di formazione per saldatori in una realtà in cui non esistono fabbriche siderurgiche significa comunque destinare quell'attività all'insuccesso per un'offerta lavorativa che sia coerente col territorio. Vi invito, quindi, a tenere presente il fatto che, se vogliamo creare corsi di formazione che portino a sbocchi lavorativi, sarebbe opportuno tener conto delle esigenze lavorative di quel territorio. dunque attenzione a quello che state facendo e dite agli italiani che volete trasbordarli lontani dalla loro terra, altrimenti perdono il reddito di inclusione.

ripetere per l'ennesima volta quello che ho spiegato in Commissione. Questo emendamento cercava di dare una mano alla maggioranza, in quanto a nostro avviso stiamo sovraccaricando i servizi sociali dei nostri territori, quindi gli assistenti sociali dei Comuni,

credo che tutti i colleghi e le colleghe sappiano che stiamo qui parlando dell'offerta congrua, e cioè di quella che dovrebbe essere un'offerta di lavoro per chi percepisce il reddito di inclusione o per chi è avviato ai corsi di formazione, che non può essere rifiutata, pena la perdita del beneficio.

che comunque, visto che l'obiettivo è sottrarre quelle persone alla povertà, ci fosse una condizione tale per cui il loro reddito e la retribuzione oraria non fosse inferiore a 9 euro lordi all'ora. È una condizione questa che non solo riconosce che il lavoro va pagato in ragione della sua qualità qualità e della quantità della prestazione, ma che serve anche a costruire un retroterra per quelle persone che permettano loro non di campare qualche tempo, ma di uscire dalla trappola della povertà e ad avere una prospettiva. Come potete vedere, è un emendamento firmato da molte delle opposizioni presenti in quest'Aula ed era un'occasione per dire che non si vogliono persone povere, lavoro povero, ma si vogliono invece dare delle risposte positive. Credo che sarebbe utile che il Governo e la relatrice ci ripensassero prima di continuare a bocciare qualunque cosa che serve a dare una prospettiva di uscita dalla povertà a chi oggi ne ha bisogno.

a me pare che dovremmo tutti pensare se davvero crediamo che un lavoratore o una lavoratrice di fronte a una proposta di lavoro, maggiormente se a lunga distanza, possa accettarlo o se debba avere delle condizioni. Negando

e di dare possibilità di lavoro, ma nei fatti impedite di accettare le proposte. È impossibile per un lavoratore di Napoli pensare di arrivare a Lecco senza avere una garanzia e una condizione almeno dignitosa dal punto di vista della retribuzione.

«Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa». questo decreto non dà tutele al lavoratore. Noi chiedevamo esclusivamente che ci fosse una tutela secondo l'articolo 36 della Costituzione,

è sicuramente importante, ma richiede una serie di competenze digitali. Non so se voi avete avuto l'occasione di parlare con chi ha percepito il reddito di cittadinanza

L'istituzione di un fondo per le competenze digitali, che costa 5 milioni di euro, va a colmare questo *gap* del disegno di legge in esame e, quindi, è migliorativo nella direzione che doveva servire proprio alla formazione del lavoro.

non possiamo non riconoscere una tale necessità che ha la popolazione che si dovrà poi fornire di strumenti per poter raggiungere questo obiettivo, che è l'agognato lavoro;

Signor Presidente, questo è un emendamento che noi consideriamo tra le priorità del decreto, perché riguarda, e ci ricorda soprattutto, una vicenda molto dolorosa, quella di Luana D'Orazio, che morì proprio a causa della insicurezza dei macchinari. Noi chiediamo al Governo, che ha avuto tanto tempo per poter verificare anche le eventuali coperture finanziarie, di lasciare questo emendamento tra i prioritari, proprio perché riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, ovviamente a partire dalle aziende private.

su questo, perché lo consideriamo davvero fondamentale, visto che, purtroppo, è cronaca quotidiana vedere troppi morti sul lavoro

in esame vuole introdurre l'insegnamento della cultura della sicurezza Stiamo tutti soffrendo perché il numero delle morti bianche, delle morti sul lavoro, sta aumentando. Istituiamo una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause delle morti sul lavoro e non vogliamo introdurre nella scuola

a riflettere su questo emendamento, che è una proposta di razionalità e di prevenzione primaria, prima che accada il danno. La cultura della sicurezza deve diventare un patrimonio di tutta la Nazione e lo può diventare solo se parte dalle scuole. Questo è quello che dice l'emendamento.

Prima abbiamo parlato di competenze digitali e le avete bocciate; poi abbiamo parlato di sicurezza sul lavoro nella scuola e l'avete bocciata. Qui si parla di una cosa che tutti fanno o che poi tutti potranno fare, se vorrete, In questo emendamento chiediamo che sia data la possibilità di disconnessione durante lo svolgimento di questo tipo di lavoro. Sappiamo benissimo che cosa significa

no. Non so in che modo sia possibile parlare di tecnologia, di *smart working* e di competenze digitali. Questo è un Governo che non ragiona con i tempi moderni.

Signor Presidente, anche questo emendamento parla di sicurezza del lavoro. È un emendamento che richiede il potenziamento della medicina del lavoro.

Ma come possiamo fare prevenzione sulla sicurezza? Questo è un decreto che parla anche di sicurezza e voi state negando la sicurezza a migliaia di cittadini.

dedicate alla sicurezza sul lavoro e anche a favore dei tanti che soffrono la perdita in ragione degli infortuni e delle morti sul lavoro. Vorremmo però cogliere l'occasione - altrimenti c'è ipocrisia nelle cose che si fanno per chiedere al Presidente del Senato di farsi promotore rispetto al Governo affinché vengano ritirati quei decreti che giusto ieri avevano deciso di abbassare il massimale che si riconosceva alle famiglie

lavoro. Non violiamo ulteriormente la loro serenità attraverso ipocrisie inutili.

inserire 5 milioni in più; se però poi si sottraggono in altri provvedimenti e in altri decreti-legge, è evidente che facciamo un gioco davvero ipocrita contro le famiglie e le persone che hanno subito infortuni sul lavoro. Chiedo anch'io al Governo che ci sia una riflessione rispetto a quello che si sta votando oggi e ad altri decreti-legge su cui si sta lavorando in maniera contraria.

quindi al Governo se c'è questa possibilità, al fine di riqualificare i lavoratori delle aree di crisi industriale.

Presidente, questo emendamento riguarda il credito d'imposta, quindi vi guardiamo in faccia e vi diciamo che stiamo parlando alle imprese e agli studi professionali, qualcosa che dovrebbe essere forse caro anche a voi della maggioranza. Vi chiediamo il credito d'imposta per l'acquisto di strumenti informatici, perché ancora una volta ritornano le problematiche legate al lavoro agile, alle competenze digitali e a tutto quello che si dovrà fare grazie alle piattaforme digitali. digitali. Non credo che questo emendamento possa essere ignorato, perché significa ignorare il presente e anche il futuro della nostra Nazione. Il credito d'imposta per gli strumenti digitali non lo volete, il lavoro agile non lo volete, competenze digitali non le volete, ma insomma che tipo di Italia esce fuori da questo decreto lavoro? Io non lo so. Vi invito veramente a rivedere la vostra posizione sul credito d'imposta, perché quello che uscirà su tutti i giornali è che voi della maggioranza

soli attori che partecipano al contratto e secondo noi questo è pericoloso. Con questi emendamenti chiediamo che vengano reinserite le causali nei contratti di lavoro a termine. Non è possibile condannare alla precarietà i nostri giovani e tutti i nostri lavoratori che verranno ricattati per pochi euro al mese. Se poi aggiungiamo che avete rifiutato anche il nostro emendamento che proponeva una soglia minima sotto la quale non si può andare di nove euro l'ora, allora vuol dire che stiamo condannando le persone a lavorare per 500 o 600 euro al mese e questo non è possibile.

interviene in un'area verso la quale il Governo e la maggioranza hanno dimostrato di essere molto sensibili, ovvero il sostegno alla maternità, alla genitorialità. Riporto l'ultimo dato disponibile dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che parla, per il 2020, di 42.000 neogenitori che abbandonano il lavoro, danno le dimissioni volontarie nel primo anno di vita del figlio, perché non sono in grado di conciliare correttamente l'attività lavorativa con le esigenze della famiglia. Il dato preoccupante è che - il 75 per cento di questo numero - 37.000 sono donne. confidando nell'attenzione che questa maggioranza ha nei confronti della natalità, vi ringrazio anticipatamente per il voto favorevole che sicuramente esprimerete, anche perché questo è un sostegno alla vostra lotta, da patrioti, alla sostituzione etnica. Quindi, mi aspetto con piacere il vostro voto favorevole.

richiede un'indennità in caso di violenza di genere per le lavoratrici autonome. Credo che tutti in quest'Aula siano sensibili al problema della violenza sulle donne.

veramente una discriminazione nei confronti delle donne tutelare solo le donne nel pubblico e non le lavoratrici autonome. Chiedo che si faccia davvero una riflessione su un tema così importante come quello della violenza sulle donne.

Per effetto del parere espresso dalla Commissione bilancio, i testi degli emendamenti 28.0.1000, 28.0.100 (testo 2), 28.0.101 e 28.0.102 (testo 2), come riformulati, risultano tutti identici.

non è per aggiungere la firma ovviamente, ma voglio chiarire che si tratta di un emendamento che ho proposto e riproposto dalla legge di bilancio. È un emendamento che tutela i fragili che sono in una condizione

In Commissione ho sottolineato chi erano i fragili e ci tengo a precisare che stiamo parlando di pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria: trapianto di organo, trapianto di cellule staminali, terapia a base di cellule T esprimenti un recettore chimerico antigenico, immunodeficienze secondarie, dialisi, insufficienza renale cronica, pregressa splenectomia, sindrome da immunodeficienza, pazienti con cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, *ictus*, diabete mellito, broncopneumopatia ostruttiva cronica, epatite cronica e obesità.

Siccome quello che sta dicendo non corrisponde al vero, si va a votare una cosa che non è al 31 dicembre, ma al 30 settembre e che va a coprire dei fondi che prima non erano indicati. 28.0.1000, 28.0.100 (testo 2), 28.0.101

Signor Presidente, desidero ringraziare la relatrice perché come Lega abbiamo presentato in Commissione questo emendamento con la scadenza per i lavoratori fragili e il rinnovo al 30 settembre 2023. Lo abbiamo ritirato perché non c'erano le coperture. Ringrazio la relatrice perché ha lavorato e il Governo perché

quei 35 giovani all'indomani della fine della pandemia, sono stati tutti licenziati.

Il Governo, in realtà, porta avanti un percorso virtuoso che è iniziato col presidente Draghi, si è consolidato nella ultima finanziaria e anche nel decreto va avanti su questo percorso, sino ad arrivare a sei-sette punti di taglio del cuneo fiscale. Certo, non è ancora sufficiente per recuperare il potere d'acquisto dei lavoratori, visto anche il taglieggiamento dell'inflazione, ma è un passo significativo. siccome noi crediamo davvero che sia un passo importante, significativo, crediamo anche che non possa essere uno *spot*, una cosa momentanea, che dura sei mesi nelle tasche delle lavoratrici e dei lavoratori. Pertanto, nell'emendamento, creiamo e proponiamo le condizioni perché anche oltre la fine di quest'anno ai lavoratori venga consolidato il taglio del cuneo fiscale. Dove prendere le risorse? Diamo un suggerimento molto facile da poter concretizzare. Noi siamo un Paese che, tra evasione fiscale ed evasione contributiva, conta circa 150 miliardi all'anno. Ecco dove trovare i 10 miliardi

il recupero, che c'è stato quest'anno, dell'evasione fiscale per restituirlo a chi le tasse le paga: i lavoratori e le lavoratrici. E magari, tutti assieme in quest'Aula, vediamo quale piano strategico importante il Governo ha per una lotta davvero importante, senza quartiere all'evasione fiscale.